Onorevoli colleghi, l'immane tragedia che sabato scorso ha colpito al cuore la Polonia suscita in tutti noi un moto di sgomento e di partecipazione al profondo dolore che ha scosso una Nazione antica e fiera, legata al nostro Paese da una profonda e secolare amicizia. La scomparsa improvvisa e drammatica, insieme al presidente Lech Kaczynski, di tanti esponenti delle istituzioni polacche - tra cui la vice presidente del Senato Krystina Bochenek, due Vice Presidenti del Sejm, tredici membri del Governo, il Governatore della Banca centrale, i vertici delle Forze armate e l'Ordinario militare di Polonia - evoca, per la seconda volta in pochi decenni, lo spettro della decimazione della classe dirigente polacca. L'aereo presidenziale precipitato era infatti diretto - come è noto - ad una cerimonia di commemorazione dell'eccidio di Katyn: in quelle oscure foreste, 70 anni or sono, le forze sovietiche sterminarono migliaia di ufficiali dell'esercito polacco, con il fine dichiarato di sopprimere l'*élite* dello Stato invaso nel 1939. Il primo a porre in relazione i due tragici eventi è stato l'ex presidente della Polonia e premio Nobel per la pace Lech Walesa, il quale ha sottolineato come mai forse, prima d'ora, la storia avesse colpito così duramente un popolo per due volte nello stesso luogo. Auspico che l'Italia e l'Europa sapranno farsi vicine, nella condivisione dei medesimi ideali di libertà e di solidarietà, al dolore della Polonia ferita, e raccogliere la preziosa testimonianza del suo impegno nel ricomporre e superare le ferite sanguinose inferte al nostro Continente dalla storia del Novecento, attraverso il difficile cammino della memoria e della riconciliazione. Uno storico segno di questo spirito è stato la scelta della Federazione russa di proclamare il lutto nazionale a seguito della tragedia, quale testimonianza tangibile di partecipazione al dolore del popolo polacco. Proprio nello spirito di vicinanza e solidarietà ora ricordato, ho ritenuto opportuno annullare la cena di gala già prevista per la serata di giovedì prossimo in occasione della XII riunione dei Senati d'Europa, che si terrà in questa città. Sono quindi certo di esprimere il sentimento dell'intera Assemblea nel rivolgere un pensiero di affettuosa solidarietà e vicinanza al collega e amico Bogdan Borusewicz, presidente del Senato polacco, ed un sentito augurio di buon lavoro al presidente del Sejm Bronislaw Komorowski, da sabato Presidente *ad interim* della Repubblica di Polonia. Invito allora tutti i colleghi ad osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento in memoria del presidente Kaczynski e di tutte le 96 vittime del disastro di Smolènsk.

In segno di lutto, sospendo la seduta per cinque minuti.

Onorevoli colleghi, come è tristemente noto a tutti voi, ieri mattina un gravissimo incidente ha coinvolto un treno regionale in Val Venosta, sulla linea tra Malles e Merano, provocando nove vittime e diversi feriti, alcuni dei quali versano, purtroppo, in condizioni molto gravi. I soccorsi, sebbene resi assai difficili dalla conformazione dei luoghi in cui è avvenuta la frana che ha provocato il deragliamento del convoglio, si sono dispiegati con grande rapidità ed efficacia: i soccorritori sono giunti a scavare con le mani nude nel fango per liberare le aperture dei vagoni e trarre in salvo le persone intrappolate al loro interno. Sono certo allora di esprimere il sentimento di tutti i colleghi nel rivolgere un commosso ringraziamento a quanti si sono prodigati nell'emergenza, dai Vigili del fuoco agli operatori della Protezione civile, dalle forze dell'ordine al personale dei servizi sanitari. Il Governo si è dichiarato disponibile a riferire all'Assemblea del Senato non appena in possesso di tutti gli elementi necessari ad una prima, esauriente risposta circa le cause e la dinamica di quello che certamente è uno dei più gravi disastri ferroviari degli ultimi anni. Già nella mattinata di ieri ho inviato al presidente della Provincia di Bolzano Luis Durnwalder un messaggio di vicinanza alle famiglie delle vittime e di affettuosa solidarietà ai numerosi feriti. Sentimenti che qui rinnovo, a nome mio personale e di tutta l'Assemblea. In segno di cordoglio per le vittime di questo grave incidente, fra le quali si contano purtroppo diversi giovani, invito i colleghi ad osservare un minuto di raccoglimento.

la terribile tragedia ferroviaria che ha colpito la Val Venosta ieri mattina alle ore 9,03 ha suscitato, nella nostra Provincia di Bolzano, sgomento e commozione. L'incidente si è verificato tra le stazioni ferroviarie di Laces e Castelbello, a 20 chilometri da Merano, sul treno regionale R108 che va da Malles a Merano. Nove persone hanno perso la vita e ventotto sono i feriti, sette dei quali in gravi condizioni. Innanzitutto, vorrei esprimere, a nome personale e a nome del mio Gruppo parlamentare, UDC, SVP, Io Sud e Autonomie, solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime e ai feriti, cui auguro una rapida guarigione. Non appena ho appreso la notizia del tragico incidente mi sono immediatamente recato sul luogo della sciagura, dato che risiedo a Silandro, che dista solo tre chilometri. Ho potuto Ho potuto constatare di persona la portata della disgrazia, che ha colpito soprattutto studenti e lavoratori pendolari. Esprimo un sentito apprezzamento per la macchina dei soccorsi, composta da circa 500 persone, tra cui i Vigili del fuoco volontari e l'Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca, nonché il Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano, il Soccorso alpino e subacqueo, i soccorritori della Protezione civile, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e la Polizia di Stato, che circa cinque minuti dopo la tragedia erano sul posto e si sono prodigati per salvare il maggior numero di persone.

che si è trattato di una tragica fatalità dovuta a un'incredibile sequenza di circostanze negative. Il dovuto ringraziamento va anche all'amministratore delegato di Trenitalia, Mauro Moretti, anch'egli precipitatosi sul posto. La mia riconoscenza va anche a lei, signor Presidente, e al Capo dello Stato Giorgio Napolitano, che ha inviato un messaggio di cordoglio. La fuoriuscita dell'acqua sul pendio a monte dei binari ha reso instabile il terreno, che improvvisamente è scivolato a valle, portandosi dietro alberi e pietre, proprio nell'istante del passaggio del treno, investendo il primo convoglio. Si è trattato di una tragica fatalità e di un incidente assolutamente imprevedibile, come evidenziato anche dal nostro presidente della Provincia di Bolzano e capo della Protezione civile locale Luis Durnwalder. Purtroppo, nonostante i sistemi di sicurezza fossero di ultima generazione, non si è riusciti ad evitare la tragedia, che ha causato tanto dolore e sofferenza tra il popolo sudtirolese, che amava questo treno pulito, sempre puntuale e che ha eliminato gli ultimi ostacoli alla mobilità delle persone diversamente abili. Auspicando un rapido chiarimento delle effettive cause della tragedia e di eventuali responsabilità, rivolgo un pensiero commosso alle famiglie delle vittime. Signor Presidente, mi unisco anch'io, a nome del Gruppo Italia dei Valori, all'espressione del più vivo cordoglio alle famiglie coinvolte nel grave incidente ferroviario e alle autorità e alle istituzioni altoatesine.

Ma è davvero pensabile che questo accada ancora nel 2010? Credo che ancora una volta torni al centro il tema della sicurezza,

specialmente in quei tratti che riguardano le ferrovie regionali e che possono sembrare secondari, ma che, come è stato già detto, interessano fortemente studenti e lavoratori,

dell'imponderabile: se quella frana fosse caduta 30 secondi prima o dopo non sarebbe successo assolutamente niente, perché i sistemi di sicurezza avrebbero bloccato la linea intera. È accaduto quello che non doveva accadere; è accaduto l'imponderabile. Ciò deve indubbiamente farci pensare che l'attenzione all'ambiente non è mai sufficiente. Io posso dire, anche a nome del collega Pinzger che proviene da quei paesi, che la Provincia di Bolzano ha fatto della gestione dell'ambiente un proprio cavallo di battaglia:

alle famiglie dei feriti la nostra vicinanza e alle famiglie delle vittime il cordoglio più affettuoso, che pensiamo possa essere pronunciato a nome di tutta l'Istituzione e di tutta l'Assemblea del Senato.

a nome del Gruppo del Partito Democratico mi associo all'espressione di cordoglio per le persone decedute nell'incidente ferroviario avvenuto lungo la linea della Val Venosta; esprimiamo altresì vicinanza alle persone ricoverate e alle famiglie delle vittime, così crudelmente provate. Con un preciso e forte colpo di maglio, la morte ha ghermito donne e uomini; le loro storie, le loro vicende personali, che abbiamo così potuto conoscere, ci hanno colpito perché immagini precise di esperienze quotidiane, di vite normali all'improvviso spezzate. In questa nostra sede istituzionale è altresì questa l'occasione di chiedere una precisa verifica delle circostanze in cui si è realizzato il disastroso incidente: ovviamente, l'esito dell'indagine aiuterà ad individuare le eventuali responsabilità. La modernità di quelle linee ferroviarie, le tecnologie applicate, la qualità dei servizi colà resi agli utenti stupiscono se confrontate con le circostanze dell'incidente. Pertanto, si pone la questione della gestione del territorio, in particolare del suolo, in quelle specifiche realtà, oggetto di una coltivazione intensiva ed organizzata. Occorrerà interrogarsi sulla necessità di accompagnare anche un utilizzo produttivo di tale qualità con una obbligatoria cura manutentiva degli impianti realizzati, che abbia altrettanta qualità e tempestività. Signor Presidente, esprimo alla collega e ai colleghi del Gruppo Südtiroler Volkspartei il rincrescimento per quelle vite perdute e, tramite loro, esprimo anche un sostegno all'azione di soccorso e agli ulteriori interventi che la Provincia autonoma di Bolzano sta impostando in queste ore per affrontare con impegno gli eventi. Grazie

Si potrebbero fare molte riflessioni - alcune sono già state avanzate - su un simile incidente, che è uguale a molti altri già accaduti anche ad altre latitudini, ma certamente in questo caso c'è un connotato che è già emerso nel dibattito, quello della vita in montagna, di chi fa la scelta di rimanere a vivere - o a sopravvivere, in certi casi - in zone impervie, dove vivere è una conquista quotidiana ed è una sfida all'ambiente, oltre che agli equilibri circostanti. Parlo anche come vice presidente vicario del gruppo parlamentare "Amici della montagna": 198 senatori e deputati che hanno inteso manifestare con questa adesione la loro attenzione, la loro particolare sensibilità per le problematiche delle zone di montagna, che non sono zone svantaggiate, come qualche volta qualcuno intende etichettarle, ma zone particolarmente sensibili. Voglio anch'io testimoniare, visto che abitando nella limitrofa Provincia di Trento conosco bene quelle realtà, il perfetto funzionamento degli apparati di soccorso e soprattutto il grande spirito di solidarietà che immediatamente si è manifestato. La montagna, purtroppo, è un ambiente affascinante, suggestivo, generoso, ma molto severo con chi lo ha scelto come *habitat*. Accanto a questa sciagura, signor Presidente, anche questa settimana, nonostante tutte le raccomandazioni e le esortazioni alla prudenza, abbiamo visto visto mietere altre vittime dalle valanghe, un'altra calamità naturale che durante tutta la stagione invernale ha falcidiato vite umane, in larga misura giovani; un altro segnale di quanto sia difficile vivere in montagna, di quanto, quindi, la montagna abbia bisogno di una solidarietà nazionale che spesso non le è stata manifestata. Rinnovo i sensi del cordoglio e anch'io, signor Presidente, la gratitudine per questa occasione che viene data di parlare di problemi reali, problemi di questo genere che accomunano comunità, magari numericamente non rilevanti (tutta la Regione Trentino-Alto Adige sfiora appena il milione di abitanti), ma che non per questo vanno considerati isolati e lontani. Grazie ancora. Onorevoli colleghi, lo scorso 11 aprile il senatore a vita Emilio Colombo ha compiuto il suo 90° compleanno. Ad un così elevato traguardo anagrafico corrispondono, come tutti sapete, oltre sessantacinque anni di ininterrotta attività politica. Giunto all'impegno politico dopo una feconda attività in seno alle associazioni cattoliche, nelle quali ricopre numerosi incarichi di responsabilità, fra cui quello di vice presidente nazionale della Gioventù italiana di Azione cattolica, a soli 26 anni diviene uno dei più giovani costituenti, eletto nella circoscrizione di Potenza e Matera. Dal 1948 al 1992 Emilio Colombo è costantemente confermato dal corpo elettorale, con larghissimo suffragio, quale membro della Camera dei deputati. Una fotografia - che so essere molto cara al presidente Colombo - lo ritrae, durante una campagna elettorale degli anni Cinquanta, a margine di un comizio nella città di Matera, mentre si intrattiene con un gruppo di cittadini e prende nota delle loro istanze. Ritengo che quell'immagine simboleggi con grande efficacia una concezione dell'attività politica che, senza distogliere l'attenzione dai grandi problemi della vita interna ed internazionale, sa trarre la sua linfa vitale dall'ascolto e dal confronto diretto con la vita concreta dei cittadini, con i loro bisogni, con le loro speranze. Un atteggiamento che è valso ad Emilio Colombo un sostegno senza eguali da parte dell'elettorato, che ha toccato il suo massimo grado nel 1979, quando, in occasione delle prime elezioni a suffragio universale del Parlamento europeo, riscosse quasi novecentomila preferenze individuali. Il 14 gennaio 2003, nominato senatore a vita dal presidente Ciampi per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale, è entrato a far parte della nostra Assemblea. Ancor più che nell'attività parlamentare, è però nell'esercizio delle funzioni di Governo che Emilio Colombo si è reso protagonista della storia politica del nostro Paese: salvo brevi periodi, pressoché tutti i Governi della Repubblica fino al 1992 lo hanno infatti annoverato tra i loro componenti di primo piano. Quando non sedette nel Consiglio dei ministri, come accadde ad esempio durante la VII legislatura, fu per ricoprire alti incarichi in ambito internazionale e comunitario, tra i quali quello di Presidente del Parlamento europeo dal 1977 al 1979. Sottosegretario all'agricoltura nel V e nel VI Governo De Gasperi, è il principale collaboratore di Antonio Segni nella preparazione e nell'attuazione della riforma agraria del 1950. Quando Segni viene incaricato di formare il suo primo Governo, nel luglio del 1955, Emilio Colombo gli succede a capo del Dicastero dell'agricoltura: è l'inizio di una straordinaria serie di incarichi ministeriali che, in particolare come titolare di Ministeri economici - quali l'industria, il tesoro, il bilancio e le finanze - tra il 1958 e il 1970, hanno reso il nostro collega protagonista di una stagione segnata dal rigore finanziario e dalla stabilità monetaria, nonché dal più grande impegno profuso nello sviluppo dell'integrazione comunitaria. Nell'agosto del 1970 Emilio Colombo riceve l'incarico di formare il Governo, che presiederà fino al febbraio del 1972: un biennio denso di importanti riforme, dall'attuazione dell'ordinamento regionale, con l'approvazione dei primi statuti ordinari, alla riforma fiscale, approvata nell'ottobre del 1971, che ancora disciplina, nel suo impianto generale, il nostro sistema tributario. Dopo l'esperienza a capo dell'Esecutivo, il senatore Colombo ritorna alla guida del Dicastero del tesoro sino al 1977, quando - come già ricordato - è eletto Presidente del Parlamento europeo. Per l'impegno profuso nell'evoluzione verso una rappresentanza piena e diretta del Parlamento europeo, quale tappa fondamentale del processo di integrazione comunitaria, viene insignito ad Aquisgrana, nel maggio del 1979 - terzo uomo politico italiano dopo Alcide De Gasperi ed Antonio Segni - del «Premio Carlo Magno», che viene assegnato ogni anno alla personalità del continente che ha maggiormente contribuito allo sviluppo delle istituzioni europee. L'impegno verso la costante crescita dell'integrazione comunitaria, insieme allo sviluppo delle istituzioni multilaterali ed al crescente dialogo tra Est ed Ovest, continuerà ad animare l'attività di Governo del senatore Colombo, nella nuova veste di titolare del Ministero degli affari esteri, incarico ricoperto in numerose compagini ministeriali dal 1980 al 1992. Anche dal suo seggio di senatore Emilio Colombo ha continuato ad esortare i colleghi parlamentari ed i Governi che si sono succeduti dal 2003 ad oggi

alla fiducia incrollabile nei destini di un'Europa forte e coesa. Sono certo perciò di interpretare l'animo di tutta l'Assemblea nel rinnovarle, senatore Colombo, i più affettuosi auguri, assieme ad un sincero ringraziamento per lo straordinario bagaglio di esperienze che lei continua a mettere a disposizione della nostra istituzione e dell'intero Paese. Grazie!

siamo qui per festeggiare i 90 anni di un grande protagonista della politica e della vita democratica del nostro Paese: i senatori dell'UDC, SVP, Io Sud e Autonomie, Gruppo parlamentare che si onora di averlo come componente, formulano i loro più affettuosi auguri di compleanno al senatore Emilio Colombo. Emilio Colombo, grazie ad una prestigiosa storia personale, può essere annoverato tra gli esponenti più significativi della storia repubblicana del nostro Paese. Nella sua lunga esperienza parlamentare, e soprattutto nei suoi diversi incarichi di governo, nazionali ed europei, che lei ha giustamente ricordato, signor Presidente, egli è riuscito a rendere patrimonio comune e condiviso una politica orientata alla crescita morale e civile dell'intero Paese. Nel 1948, all'età di soli 26 anni, è eletto deputato alla Costituente nella circoscrizione di Potenza-Matera, e siede in Parlamento per numerose legislature, ricoprendo, tra le altre, le cariche di Ministro delle finanze, del tesoro e degli affari È per due volte Presidente del Consiglio dei ministri e, grazie al suo impegno europeista, nel 1977 è eletto Presidente del Parlamento europeo. Emilio Colombo è l'uomo politico che ha contribuito in maniera determinante alla ricostruzione del Paese nel dopoguerra, ed è stato anche un indiscusso protagonista all'interno della Democrazia cristiana, iniziando la sua carriera politica da giovanissimo nell'associazionismo cattolico, e in particolare nell'Azione cattolica. La politica italiana ed internazionale lo ha visto protagonista: la sua è una politica basata sull'etica dell'ascolto e soprattutto sull'esigenza del confronto umano, fondata sull'impegno sociale non generico né distaccato. Una politica, quella di Colombo, che ha attraversato tutta la storia dell'Italia dal dopoguerra ad oggi, impegnata per la crescita morale e civile del Paese, per la valorizzazione dei suoi territori e delle sue ricchezze. Tutti principi, questi, a cui noi dovremmo rivolgerci, specialmente in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo oggi: un periodo di crisi e di incomprensioni, dove il conflitto, soprattutto in politica, vince sul dialogo. E come ha ricordato il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Emilio Colombo è stato al servizio di questo Paese, sempre nel segno della fedeltà ai principi costituzionali ed alle istituzioni repubblicane. Ha raggiunto il traguardo dei 90 anni con intatta forza ideale e morale e con sempre serena determinazione nel perseguire il bene comune. Per questi motivi il presidente Colombo è, e deve essere, un esempio per noi: come strenuo difensore dei principi costituzionali e della Repubblica democratica parlamentare. Quei principi che oggi sembrano, a volte, obsoleti sono invece la base del funzionamento regolare della vita democratica di un Paese. Bisogna, quindi, andarci piano quando si parla di riforme e soprattutto non bisogna farsi prendere da una schizofrenia in questo senso. Le riforme vanno fatte, ma dobbiamo evitare, come dice il presidente Colombo «le tendenze plebiscitarie, autoritarie, e la forte accentuazione del personalismo». Facendo sempre riferimento anche alla vita democratica all'interno dei partiti, il presidente Colombo ha sottolineato questo aspetto: «Non si capisce che le future classi dirigenti si formano nei partiti. E che i partiti, quelli veri, sono necessari». Nel corso degli innumerevoli incarichi ricoperti, egli ha sempre mantenuto altissimo il suo senso dello Stato e conseguentemente si è comportato da uomo di Stato, dando un'ottima immagine dell'Italia all'estero. se, nella lunga e straordinaria attività svolta da Emilio Colombo, volessimo andare alla ricerca degli elementi in grado di sintetizzare la natura del suo impegno e la qualità del suo servizio alle istituzioni, non potremmo che pensare innanzitutto ai temi dell'unità europea e dello sviluppo del Mezzogiorno. Due riferimenti costanti che lo hanno accompagnato nel difficile cammino dall'Assemblea costituente ad oggi. Dal lodo di Melissa alla riforma agraria e alla Cassa per il Mezzogiorno, dai Trattati di Roma alla stagione costituente dell'Unione. Dalla diretta esperienza della Basilicata del dopoguerra ha tratto la spinta ad assumere il riscatto del Mezzogiorno non solo come importante eredità delle pregevoli analisi e proposte dei meridionalisti di fine Ottocento e del primo Novecento, ma come sfida con la quale misurarsi concretamente. Come ebbe a sottolineare, ad esempio, nel discorso pronunciato all'inaugurazione della Fiera del Levante nel 1970 da Presidente del Consiglio: «non "uno" dei problemi italiani, ma "il" problema dell'ordinato sviluppo del Paese». Lo aveva sostenuto con forza già nel 1954 al Congresso nazionale della DC di Napoli, con un discorso memorabile con il quale difese e rilanciò la strategia riformatrice dei Governi De Gasperi, giudicandola come «lo strumento di rottura di un vecchio equilibrio cristallizzato per intraprendere il colloquio con ceti fino ad oggi esclusi dal ciclo della vita democratica». Negli anni successivi sostenne con convinzione le azioni volte a favorire il processo di diffusione territoriale delle industrie, convinto che fosse «nell'interesse dell'economia nazionale e meridionale che l'industrializzazione non si risolvesse in una concentrazione di impianti in pochi centri». Aree industriali, incentivi fiscali e finanziari, infrastrutture dei territori, sostegno agli investimenti, sviluppo delle piccole imprese, finalizzazione del credito, contrattazione programmata e così via; tante tessere di un mosaico che documenta un'attenzione costante ed una particolare attitudine alla concretezza operativa. La stessa che costella anche il suo impegno per l'Europa, mai fumoso o retorico, ma fatto di gesti, di atti e di scelte. Quelle che lo hanno portato in quest'Aula oggi, a novant'anni, interprete e testimone della storia e al tempo stesso anche attore della politica, quella con la "P" maiuscola. Grazie e tanti auguri, presidente Colombo! Presidente Schifani, colleghi, ho davvero il piacere di porgere ad Emilio Colombo i migliori auguri per i novant'anni che ha recentemente compiuto, e lo faccio a nome mio personale e di tutto il Gruppo dell'Italia dei Valori. Questa lieta ricorrenza merita da parte mia poche, brevi, ma sincere riflessioni, per non indulgere in retoriche affermazioni, che questa circostanza certo non merita. Quando da giovane ginnasiale la mia famiglia si trasferì nella città natale di Emilio Colombo non avrei mai pensato di poter un giorno sedere insieme a lui tra i banchi severi e ricchi di memoria di Palazzo Madama. La sua storia istituzionale e i suoi prestigiosi incarichi, già all'epoca particolarmente importanti, facevano da contraltare ai cambiamenti che avvenivano tumultuosi in Europa e nel mondo alla fine degli anni '60. Costituente, numerose volte Ministro, Presidente del Consiglio dei ministri e del Parlamento europeo, punto di riferimento del cattolicesimo democratico, Emilio Colombo ha sempre cercato la sintesi virtuosa tra gli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa e la laicità dello Stato, che per lunghi tratti di tempo è stato elemento caratterizzante della vita politica e sociale del nostro Paese, così come proprio l'Assemblea costituente aveva voluto (laicità dello Stato di cui oggi purtroppo si stanno perdendo le tracce), in uno con gli insegnamenti dei Padri della Patria. D'altra parte, la sua partecipazione ai lavori per la nostra Costituzione rafforzò in Emilio Colombo la consapevolezza della centralità del Parlamento per il rafforzamento della libertà e della democrazia nel nostro Paese, e questo suo condiviso convincimento egli ha espresso anche di recente in quest'Aula. La sua storia di statista ha lasciato una traccia profonda in Italia, in Europa e nella tua, Presidente Colombo, nella nostra terra di Basilicata. Auguri ancora, presidente Colombo, e grazie per il tuo impegno permanente per la nostra Italia. Signor Presidente, colleghi, anch'io, a nome del Gruppo Misto, il Gruppo di cui il presidente Colombo faceva parte fino a qualche anno fa, sento il dovere di fargli gli auguri

la prima volta alla Costituente, credo ci ricordi quello spirito costituente che animò i Padri fondatori della Repubblica. In questo periodo in cui spesso qualcuno parla anche di riformismo velleitario, ritengo che un insegnamento del genere, con l'Assemblea costituente che negli anni 1946-1947 vide il cattolicesimo popolare, i liberali, il socialismo stare insieme intorno a un tavolo e dare la Carta costituente al Paese, Paese, e questa presenza ci invitino ancora una volta a recuperare questo spirito unitario: altrimenti, non andremo da nessuna parte. Se saremo insieme e uniti, se faremo le giuste mediazioni tra le diverse culture, credo che riproporremo al Paese ancora una volta la storia della prima

anche ai momenti di crisi della Democrazia cristiana. Nel 1994, dopo Tangentopoli, ha partecipato al cambiamento e alla trasformazione di quel partito nel Partito popolare.

spesso ci ricorda - ma affermando i diritti di un popolo che la storia ha penalizzato da 150 anni a questa parte, per poter tutti, come classe

città (capoluogo del Molise), quale è Campobasso, lei ha inaugurato, insieme a Papa Giovanni Paolo II, un centro di ricerca che oggi potrebbe rappresentare un'idea vincente delle nostre Regioni che inseguono il progresso.

utili alla storia del proprio Paese. Auguri di nuovo, presidente Signor Presidente, se cercassimo nell'Aula del Senato una personalità che rappresenti i due pilastri fondamentali della proiezione internazionale dell'Italia, ovvero l'idea europea e l'Alleanza atlantica, non vi sarebbe - - e non vi è - altra figura in grado di rappresentarli e di testimoniarli con altrettanta coerenza e chiarezza quanto il senatore Emilio Colombo. Colombo è stato uno degli elementi portanti di decenni di politica estera nazionale e dell'affascinante e faticoso cammino dell'integrazione dell'Italia in Europa. Come lei ha ricordato, signor Presidente, è stato tra i dirigenti politici nazionali di primo piano che non hanno avuto timore ad occuparsi dell'Europa, in stagioni nelle quali, purtroppo, un certo provincialismo delle classi dirigenti spingeva a scegliere poltrone nazionali piuttosto che un impegno nell'orizzonte di quella che era la nascente Comunità. Colombo è stato un uomo di Stato e il suo bilancio - cito solo l'esperienza da Ministro delle finanze - resta come una delle pagine più lineari e convincenti di quella stagione politica e di governo. Mi sia consentito però ricordare, colleghi, nella vita e nell'esperienza politica di questo uomo il rapporto con la sua Basilicata.

dipingere, ne «Il Vangelo secondo Matteo», l'estrema arretratezza tale da far assomigliare i sassi di Matera alla Gerusalemme dell'età di Cristo, lo si deve a classi dirigenti che hanno creato un differenziale di sviluppo in Basilicata che, da una parte, ha tenuto lontano dagli spazi della vita pubblica l'infiltrazione criminale e mafiosa e, dall'altra, ha permesso un incontro fertile e non infecondo, come in altre circostanze si è determinato, tra gli eredi delle culture democratiche principali della nostra Repubblica. tratta di un'esperienza che ancora vive e che ha bisogno certamente di aggiornamenti, ma la si deve in misura molto significativa all'equilibrio, alla capacità di innovazione e all'amore per la sua terra che il senatore Colombo ha saputo nutrire. È stato, signor Presidente, un atto di civiltà e di responsabilità da parte di Emilio Colombo il rammarico che ha rivolto in pubblico nei giorni scorsi per una vicenda personale che lo ha toccato. Non poteva mancare in queste giornate. L'ha assicurato con appropriatezza e dignità. signor Presidente, la sua testimonianza politica. A novant'anni è - a mio modo di vedere - l'esercizio ineccepibile del mandato di senatore a vita.

almeno oggi si potrà dire, in occasione della festa di compleanno del presidente Colombo, che c'è un modo di interpretare il mandato di senatore a vita che non è né fazioso né anodino. Non potrebbe che essere così. Chi può vantare un tale *cursus* istituzionale non può e non deve essere partigiano, né può nascondere i valori cui si è ispirato in tutta la sua vita politica, per primi - nel caso del presidente Colombo - quelli di un cristiano in politica quelli di un'esperienza cristiano-democratica che al compiersi dei novant'anni mantiene tutta la chiarezza e la solidità di ispirazione. Proprio di questo, nell'Aula del Senato, lo ringraziamo: dell'esercizio della qualità di senatore a vita al quale certamente i lavori di quest'Aula possono ispirarsi e dal quale possono ricavare un motivo di riconoscenza oltre che l'espressione di un augurio sincero.

riflette un ideale di politica basato sull'etica dell'ascolto ma anche sull'esigenza di un confronto umano, un impegno sociale non generico né distaccato. Nella riforma agraria, ad esempio, così come nel recupero dei Sassi di Matera, la politica impegnata per la crescita morale e civile della popolazione e per la valorizzazione rispettosa del territorio e delle sue ricchezze ha trovato una esemplare sintesi dei suoi ideali e dei suoi metodi. Il presidente Colombo può considerarsi un politico del Sud che può contare ancora su un consenso popolare incredibilmente vasto, specialmente tra gli agricoltori della sua Lucania. Il presidente Schifani e tutti i colleghi che mi hanno preceduto hanno già tracciato le tappe di un percorso politico straordinario che, come tutti hanno ricordato, nasce nel 1946, quando il presidente Colombo, a soli 26 anni, è stato eletto deputato all'Assemblea costituente. Emilio Colombo non è sicuramente uno spettatore, ma un attore della politica di questo Paese dal dopoguerra ad oggi.

porgere gli auguri al presidente Emilio Colombo e di esprimere gratitudine a quella scuola politica che ha consentito anche a me di arrivare fin qui e di farlo nel PD, ancora con lui. Noi eravamo insieme nella DC e siamo oggi insieme nel PD. Emilio Colombo, come molti di coloro che hanno attivamente dedicato l'attività politica militante a costruire il Paese, non solo a ricostruirne dalle macerie le strutture e le istituzioni, fu «inviato» nell'agone politico dai suoi educatori. Nella DC era abbastanza naturale assumere ruoli politici e sottoporsi al vaglio elettorale provenendo dall'associazionismo cattolico, dalla università cattolica, dall'Azione cattolica, dagli oratori, cioè da quegli ambienti dove non si faceva scuola politica ma si allenavano le persone ad essere cittadini, ad affinare i talenti e a mettersi a disposizione della comunità civile. È la scuola che gli ha consentito di mantenere intatta per tutta la vita, sempre, una invidiabile onestà intellettuale. I tempi del nostro amico senatore a vita ci riportano, infatti, lontano nel tempo, agli anni della Costituente di cui fu giovane deputato. Colombo ci offre l'occasione per una riflessione su una lunga stagione politica, che ha visto prima affermarsi il partito della Democrazia cristiana, poi la sua eclisse e, infine, la sua scomparsa con la nuova presenza di frammenti di successione in movimenti diversi. però, perché per i più anziani può esservi un ricordo ancora più antico e, per certi versi, più denso di evocazioni politiche e culturali, con riguardo al Colombo che era un dirigente centrale dell'Azione cattolica ed esprimeva una tendenza al rinnovamento del Paese che si innestava, nel processo di ricostruzione del dopoguerra, nella sezione più giovane e promettente della squadra di Alcide De Gasperi. Emilio Colombo non è stato un tecnico specialistico a senso unico e, quindi, unilaterale: abbiamo incontrato, in primo luogo, come esponente del movimento cattolico italiano, non solo partitico, ma di quello che si nutriva dell'insegnamento sociale della Chiesa cui fare riferimento per l'azione politica. Poi lo abbiamo trovato come una delle guide della vita economica del Paese, come Ministro di vari Dicasteri economici o con un forte impatto economico. Ha svolto anche importanti ruoli culturali, che sono stati tutti citati e sui quali non ritornerò. è stato anche presidente dell'Istituto Toniolo, quello che ha promosso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e di Roma. È un periodo lungo, si potrebbe parlare di un secolo quasi intero di storia politica e istituzionale che ha visto sempre presente e attivo Colombo: come Ministro, come Presidente del Consiglio, come figura eminente del Parlamento europeo, di cui fu presidente per tre turni. Più di altro ha segnato l'azione di Emilio Colombo la sua visione di politica estera, in cui ha svolto ruoli importanti fino alle ultime conferme della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, quando toccò a lui convincere i sovietici a non mollare l'impresa alla quale, in fondo, avevano dato anch'essi un forte contributo. La dimensione europea emerge nella vita di Colombo quasi come un presupposto non solo di una cultura politica, ma di una cultura complessiva. Un tema che si è legato e continua a legarsi all'idea di uno scenario di pace e di collaborazione tra i popoli, in cui i cattolici democratici si sono impegnati con successo per decenni. La generazione alla quale appartiene Colombo ha elaborato una costruzione democratica che appare distanziarsi dalle costruzioni spesso effimere degli epigoni di oggi, che sembrano gestire più di quanto non sia avvenuto nel passato la vicenda del momento, in un riformismo senza una prospettiva di ordine nuovo. Oggi dobbiamo riconoscere che si deve a persone come Colombo un agire per niente ripetitivo. La sua azione (come quella di quanti hanno dedicato la loro vita ad un'attività politica concepita come missione), anche se segnata dagli anni, porta un patrimonio di valori che viene dagli insegnamenti di Camaldoli, dalla teologia delle realtà terrene, di Maritain e di altri. L'attività politica di Colombo non piaceva alla sinistra democristiana nella quale io militavo. Però era una politica che, vista a distanza di tempo, appare nelle sue strutture unitarie e nella comunanza di una fede nell'impegno temporale. La rievocazione, come tutte le rievocazioni, serve a questo: a renderci ancora presente un passato in cui ci si riconosce non solo come memoria, ma anche come esperienza politica significativa, con una visione delle istituzioni e dei rapporti politici anche tra maggioranza e opposizioni che non solo solo meritano rispetto postumo, ma anche un'attenzione di esemplarità. Contrariamente ad altri amici della medesima generazione, Emilio Colombo non ci ha ancora affidato per iscritto i suoi ricordi, che non sono aneddoti personali, ma spezzoni di vita nazionale. Lo invito ancora a scrivere. Non può non lasciare testimonianze importanti. Se decidesse di dedicarvisi sarebbe non un dono alla storiografia, bensì una testimonianza di grande momento. Certamente, i primi novant'anni di una persona si celebrano con un misto di rimpianto e di nostalgia, ma anche di speranza per un futuro che ci auguriamo tutti che continui, non solo per dare un lustro permanente alla Repubblica, ma anche contributi di conoscenza e di esperienza che oggi sembrano mancare in modo deplorevole. Auguri dunque, presidente Colombo, e grazie per quanto ha già fatto per il Paese, nella speranza che rimanga un segno pedagogico per chi ci seguirà:

devo alla sua cortesia se posso, in deroga all'organizzazione consueta dei lavori e in occasione dei novant'anni del presidente Colombo, dar voce ad un sentimento di ammirazione, di gratitudine e di amicizia verso colui che considero un maestro della mia formazione politica nella Democrazia cristiana e nella mia intera esperienza nelle istituzioni. Desidero, presidente Colombo, confermarle ammirazione per la sua dirittura, per lo spessore della sua testimonianza, per il servizio verso l'Italia e l'Europa; gratitudine per tutto ciò che ci ha trasmesso in termini di valori in tempi cosi difficili e controversi; amicizia per l'apertura umana, intellettuale e morale che ha riservato ad intere generazioni. Lei ci ha insegnato che una delle missioni più alte della politica sta nell'offrire al Paese la testimonianza di come si possano conciliare interessi e valori, di come sia centrale il perseguimento del bene comune e di come le prospettive di un Mezzogiorno virtuosamente governato coincidano con quelle di un'Italia unita proiettata in Europa e nel mondo con la ricchezza delle sue risorse naturali e civili. ci ha insegnato anche che fra conservazioni ed estremismi vi è uno spazio di realismo e di sapienza che costituisce la garanzia di un ordine civile ed avanzato, nel quale trovano risposte libertà e sicurezza, diritti e doveri, lavoro, sviluppo e legalità. Continui ad offrirci il suo contributo, presidente Colombo, e continui a guidarci in questa complessa stagione, ad illuminarci con la sua lucida ed esigente intelligenza, a credere nel valore delle istituzioni e nel Parlamento come cuore pulsante di una grande democrazia. È questo il dono più prezioso al quale aspiriamo. Auguri, presidente Colombo! Signor Presidente, onorevoli colleghi, si è scritto che da buon meridionale il senatore Emilio Colombo non gradisce essere celebrato, neppure nel giorno del suo 90° compleanno. Non ama essere celebrato, ma preferisce offrire spunti di riflessione. In questo senso proverò brevemente a sottolineare qualche tratto della sua lunga e prestigiosa esperienza politica ed istituzionale per trarre qualche riflessione per il presente. Intanto, è bene sottolineare che è figlio di una piccola ed orgogliosa terra, dell'unica Regione che si può permettere di avere due appellativi - Basilicata e Lucania e che, seppur piccola, ha due versanti, bagnati da due mari: il metapontino, che affaccia sul mare Ionio, e quello della perla di Maratea, sul Tirreno. Si racconta che i Romani durante l'Impero, per piegare la fierezza di questo piccolo popolo, non incline alla sottomissione, lo esclusero dalle grandi vie di comunicazione, e quella terra pagò per secoli il prezzo dell'isolamento. questo popolo per anni andò fiero di Emilio Colombo: il suo itinerario politico rappresentò una sorta di riscatto di una Regione che negli anni successivi al secondo conflitto mondiale viveva la piaga della miseria, della povertà, dell'analfabetismo, delle grandi ondate migratorie, come documentano l'inchiesta parlamentare degli anni Cinquanta presieduta dall'onorevole Ambrico ed i rapporti sulla visita di De Gasperi

Colombo legò la sua battaglia politica a questi grandi temi sociali che entrarono di forza nell'agenda dei primi Governi repubblicani. La riforma agraria La riforma agraria trasformò in tutto il Mezzogiorno il latifondo improduttivo in una rete di poderi produttivi, assegnando campi ed abitazione a braccianti senza terra, sottratti così alla fame ed all'indigenza. Si ricorda che nel 1948 De Gasperi e Segni lo inviarono - all'epoca giovane Sottosegretario di Stato per l'agricoltura - a Melissa, in Calabria, per tentare una difficile mediazione in un aspro conflitto sociale che si era aperto proprio per l'occupazione delle terre. La mediazione gli riuscì, e questa opera gli valse come viatico per il suo cammino istituzionale. La legge sui Sassi di Matera trasformò gradualmente quella vergogna nazionale in patrimonio mondiale dell'umanità, riconosciuto dall'UNESCO, con un contestuale programma di edilizia sociale per il trasferimento delle famiglie che prima vivevano nei Sassi, progetti su cui lavorarono grandi urbanisti come Luigi Piccinato e Ludovico Quaroni. L'industrializzazione degli anni Sessanta, con l'inizio dello sfruttamento dei primi giacimenti metaniferi, diede vita ai primi poli industriali della chimica, con il coinvolgimento dell'ENI di Enrico Mattei. La prima grande infrastrutturazione viaria e la progettazione e realizzazione degli schemi idrici affrontarono, con il sostegno della Cassa del Mezzogiorno, le problematiche dell'isolamento e dell'accumulo e della distribuzione delle risorse idriche, come presupposti per dare impulso a nuove dinamiche di sviluppo. Emilio Colombo ha goduto fino agli anni Novanta di un rapporto con il suo popolo che con linguaggio odierno potremmo definire plebiscitario

nella circoscrizione meridionale per la prima elezione diretta del Parlamento europeo. Egli rappresentava l'emblema di una generazione di cattolici che, nel dopoguerra, scelsero l'impegno politico ed istituzionale come frontiera di una testimonianza laica

monsignor Augusto Bertazzoni, vescovo lombardo, amico di don Orione, che si distinse per il suo apostolato intenso e profetico nel Mezzogiorno; monsignor Delle Nocche, altro grande vescovo che ha lasciato traccia indelebile delle sue opere sociali ed educative in terra lucana; don Giuseppe De Luca, prete lucano e romano, nel senso teologico, fortemente impegnato nelle battaglie contro il modernismo, del quale però seppe cogliere il valore di reazione ad un cattolicesimo debilitato ed incapace di reggere il confronto con il mondo moderno. Maestri che Emilio Colombo ebbe la fortuna di incontrare e che segnarono la sua vita e quella di tante altre persone meno note che pure determinarono il clima culturale e sociale di quegli anni di rinascita. Una storia che ha coinvolto diverse generazioni di amministratori su cui Emilio Colombo ha esercitato per anni carisma e guida; una trama che dopo il 1994 non è scampata alla diaspora che ha colpito l'unità politica dei cattolici italiani e che in Basilicata ha prodotto posizioni ed esiti controversi su cui sarebbe utile riflettere. Ma oggi, con austerità, presidente Colombo, festeggiamo i suoi 90 anni: una vita spesa prevalentemente a servizio degli interessi della Nazione e della sua gente. Il tempo della vita è fatto di momenti di tempo, di gloria e di errori che segnano l'esperienza di ciascun uomo, metafora del limite che ci caratterizza, contro ogni superbia ed albagia. Al presidente Colombo è capitato di vivere, anche da Padre costituente, un tempo di costruzione e di rigenerazione del Paese e del mondo, di incontrare grandi maestri e di vivere a fianco dei grandi protagonisti della politica italiana e di quella internazionale. La sua generazione porta il merito di aver ancorato l'Italia ad un sicuro assetto democratico e ad una sponda di libertà allora per niente scontata.

Il Gruppo parlamentare del PdL, a mio tramite, le formula gli auguri più sinceri nel giorno del suo 90° compleanno e si associa ai sentimenti di riconoscenza espressi dal Presidente del Senato e dall'intera Assemblea. *(Applausi).*

comincerò questo mio breve discorso in modo irrituale rispetto all'argomento

quelli che hanno voluto - e li ringrazio - intervenire in Assemblea e quelli con cui personalmente mi sono incontrato. Non saprei dire quali e quanti sentimenti si affollino nel mio animo in questo momento. Innanzitutto un sentimento di gratitudine per aver voluto ricordare il senso di una lunga esperienza, da me vissuta nelle istituzioni, nel segno di un'ispirazione cristiana, che è stata essenziale nella mia visione politica.

e anche condividere il valore che ho attribuito alle istituzioni democratiche e alla centralità del Parlamento - come ha detto lei, signor Presidente, all'inizio di questo nostro incontro

i fermenti liberi e civili di una grande Nazione democratica quale è l'Italia. Ricordo ancora oggi con emozione profonda il mio primo ingresso nell'Aula parlamentare all'epoca della Costituente, nel 1946. Venivo da una combattuta campagna elettorale, che mi aveva posto di fronte a Francesco Saverio Nitti a Guido Dorso, a Carlo Levi, a Fausto Gullo, prima, e anche a Giorgio Amendola, più tardi, ed entravo in una grande Assemblea di eletti, tra i quali De Gasperi, Vittorio Emanuele Orlando, Moro, Segni, Dossetti, Fanfani, Calamandrei, Togliatti, Nenni, Terracini, Concetto Marchesi, Benedetto Croce: misurate la differenza! Credo che mai più si sia determinata nella vita democratica italiana una così fitta e preziosa confluenza di passioni politiche e di intelligenze, regolata da un'aura di rispetto e di partecipazione ad un'altissima impresa quale è stata l'edificazione - come la definì Giorgio La Pira dell'architettura costituzionale del Paese. Oggi, se mi guardo indietro, sento l'orgoglio di essere stato parte, nelle mie proporzioni, di una pagina straordinaria della vita italiana e di averla vissuta in Italia, in Europa, nel mondo con il privilegio di rivestire responsabilità pubbliche, per le quali sono grato al mio Paese, alla gente lucana, alla Democrazia Cristiana, che mi hanno onorato di un mandato, che ho cercato di assolvere in tranquilla e consapevole coscienza. Posso dire solo che non è mai venuta meno in me, e voglio riaffermarlo qui in questa sede, la consapevolezza del limite nelle azioni di governo e della politica e che il principio di «non appagamento» mi ha sempre sollecitato a dare il meglio della mia attitudine e delle mie capacità. A 90 anni, nel tempo dei consuntivi, ringrazio tutti quanti hanno inteso rispettare e condividere il mio impegno, riconoscere la bontà delle mie intenzioni, l'onestà intransigente delle mie convinzioni e perdonare le mie impazienze e gli errori di cui è lastricata la strada di ciascuno di noi. Se c'è un messaggio che vorrei affidare a chi è più giovane di me, a quanti sono, per fortuna, tanto giovani, benché senatori in quest'Aula, è di credere nella democrazia senza imboccare scorciatoie, di difenderla dalle tossine del populismo

se persuade che la democrazia non implichi fatica, sacrifici e coerenza. Credere nella democrazia e nelle sue istituzioni è stato per me un imperativo ancora più esigente quando, nella mia lunga esperienza, essa è apparsa minacciata e sottoposta a prove difficili. Perciò considero questa la premessa di ogni politica, un modo per difendere l'unità del Paese a 150 anni dalla sua fondazione, un modo per tenere viva una speranza civile, l'idea di un Paese che vuole continuare ad essere forte e rispettato nel mondo.

dopo averci esortato a evitare un voto poco meditato - sono le sue parole - e perciò

Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pomeriggio, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 22 aprile. aprile. Oggi pomeriggio inizierà la discussione delle mozioni sui fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione e in materia di politica ambientale. Le votazioni su entrambe avranno luogo domani. La 5a Commissione permanente è autorizzata a convocarsi oggi pomeriggio, anche in concomitanza con i lavori dell'Aula, per rendere il proprio parere sul disegno di legge di ratifica della Convenzione sulla tratta di esseri umani e sui relativi emendamenti. L'esame della predetta ratifica riprenderà in Assemblea domani, dopo il voto delle mozioni. Seguirà, sempre nella giornata di domani, la discussione delle altre ratifiche concluse in sede referente, a cominciare da quella sulla protezione degli animali da compagnia. Inoltre, nel corso di questa settimana inizierà la discussione generale sul disegno di legge di riforma della professione forense. La replica del Ministro della giustizia avrà luogo la prossima settimana, presumibilmente nella seduta pomeridiana di martedì 20 aprile. Il termine per la presentazione degli emendamenti, già previsto per questa sera alle ore 19, è stato differito alle ore 18 di venerdì 16 aprile. Il calendario della prossima settimana, oltre al seguito della riforma della professione forense, prevede poi ratifiche di accordi internazionali e documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Nella seduta pomeridiana di giovedì 22 aprile, alle ore 16, si svolgeranno, con trasmissione diretta televisiva per la durata di un'ora, interrogazioni a risposta immediata. Uno degli argomenti richiesti dai Gruppi concerne il Piano nazionale per l'infanzia e 1'adolescenza. Con riferimento al *question time* i Capigruppo hanno convenuto sull'opportunità di avviare una riflessione per rivedere le modalità di svolgimento di tale istituto di sindacato ispettivo.

la relazione del Procuratore generale della Corte dei conti, svolta in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario in data che: «Il Ministero dell'Interno, i Comandi generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno denunciato nel solo periodo gennaio-novembre 2009 221 reati di corruzione, 219 reati di concussione e 1.714 reati di abuso di ufficio. Inoltre, l'analisi dei dati operata dalla Guardia di finanza evidenzia un deciso aumento delle denunzie per fatti di corruzione e concussione accertati nel 2009, rispettivamente un

del fenomeno della corruzione nel nostro Paese, implementato dalla particolare forma di corruzione e concussione che riguarda le frodi comunitarie. Siamo giunti ad un valore accertato, è oggetto di citazione innanzi alla Corte dei conti, di 136 milioni di euro, a fronte dei 67 milioni di euro nel 2008. Le Regioni che più delle altre manifestano questa inclinazione alla crescita esponenziale sono la Lombardia, la Sicilia, il Lazio e la Puglia. Purtroppo,

sullo sviluppo del Paese in quanto tali fenomeni si verificano nell'ambito di gare di appalti, di realizzazione di opere pubbliche e lavori, di interventi di manutenzioni su beni della collettività. Questo aumento dei fenomeni corruttivi determina un grave allarme: non è un caso che il Governo nella seduta del 25 febbraio di quest'anno, in

Il fenomeno della corruzione sta infettando, più che nel passato, la pubblica amministrazione,

costituendo la corruzione una vera e propria tassa immorale ed occulta pagata con i soldi prelevati dalle tasche dei cittadini contribuenti.

subito dopo la Turchia e a pari merito con l'Arabia Saudita. Il Consiglio d'Europa nell'ottobre 2009 ha dichiarato molto seria la situazione italiana. A fronte di questo scenario pesante ed inquietante, nel nostro Paese si è proceduto nel 2008 alla soppressione dell'Alto Commissario per la prevenzione ed ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, e alla sua sostituzione con un altro organo che, allo stato, non pare abbia ottimizzato il lavoro ed i risultati. Nella relazione presentata al Parlamento il 17 novembre 2009 è scritto: «Negli ultimi cinque anni, in tema di reati contro la pubblica amministrazione il problema centrale, prioritario, è quello di un rilevante numero di delinquenti, più o meno organizzati, che hanno scambiato la pubblica amministrazione per una sorta di bancomat senza *plafond*. Oltre il 40 per cento dei reati contro la pubblica amministrazione degli ultimi cinque anni riguardano, indebite percezioni di fondi e finanziamenti pubblici o truffe aggravate per la percezione di questi contributi: sono reati commessi da privati, che approfittano di una pubblica amministrazione senza antifurti, senza sistemi di difesa, analogamente a quanto fanno i ladri che scelgono gli obiettivi più facili». Uno degli aspetti gravi che è stato evidenziato dalla Guardia di finanza è il cambio di modalità nella confezione del reato di corruzione. Rispetto al modello classico (la *datio* del denaro *brevi manu*), oggi i corruttori costituiscono provviste di denaro mediante l'utilizzo di sovrafatturazione di operazioni commerciali e di fatturazioni di operazioni inesistenti, in ciò avvantaggiati anche dal fatto che nel nostro ordinamento è stata inserita la soglia di punibilità dell'1 per cento per il reato di falso in bilancio; sicché un'impresa con un patrimonio di 100 milioni di euro può costituire attraverso un falso un fondo nero di un milione di euro senza per ciò essere punibile. La creazione del fondo nero poi facilita il versamento di dazioni corruttive. In tutto questo si notano anche delle gravi lacune del nostro Paese: uno dei sistemi individuati, quello di obbligare le imprese appaltatrici di lavori pubblici ad utilizzare conti dedicati e a rendere possibile la tracciabilità dei flussi, purtroppo non è stato attuato. Prendiamo l'esempio del decreto per l'Abruzzo: dopo il terremoto dell'Aquila, entro il 28 maggio del 2009 doveva prevedersi la disciplina sulla tracciabilità, ma non è stato ancora fatto e non è stato fatto neanche per il decreto per l'Expo 2015. Il ministro Maroni, pochi giorni fa, in Commissione antimafia ci ha annunciato che ci sono grandi difficoltà nell'approntare il sistema di controllo dei flussi finanziari. Questo è un gravissimo problema con il quale dobbiamo confrontarci: com'è possibile che esistano difficoltà per controllare i flussi? La nostra mozione sollecita il Governo a facilitare l'approvazione dei disegni di legge

nel reato di estorsione, e la concussione per induzione facendone un'ipotesi aggravata della corruzione, superando ciò che costituisce un'anomalia ossia la scappatoia della concussione per proteggere i corruttori. Dobbiamo prevedere una disciplina che, pur prevedendo aggravanti di pena per i percettori indebiti di prezzo corruttivo, comunque non assolva il privato che facilita la sua attività pagando il pubblico funzionario. il voto in Aula di questi disegni di legge.

Onorevole Presidente, ho premuto il cronometro dei dieci minuti che mi sono assegnati e le confesso che, contrariamente al mio viziaccio di parlare a braccio, avevo preso talmente sul serio l'argomento che mi ero preparato quasi una scaletta. Poiché il Senato complessivamente non dimostra il massimo dell'interesse e del *pathos* nell'affrontare questo argomento, a braccio, sostanzialmente per dire che, se le istituzioni non prendono atto (e i partecipi delle istituzioni, quali noi siamo) che la questione morale (o questione etica, se preferite un sinonimo) torna ad essere prepotentemente centrale nel dibattito istituzionale e politico, significa che rischiamo di perdere il contatto con la pubblica opinione in maniera più drammatica di quanto mai in passato sia avvenuto. L'etica pubblica torna ad essere centrale nella conquista o nella riconquista della credibilità delle istituzioni, della politica e di chiunque sia a trattare pubblici interessi nella coscienza dell'opinione pubblica; credibilità che ha dei risvolti quali sono stati quelli dell'astensionismo nel recente turno elettorale, di cui tutti scrivono e parlano senza prendere atto del grido silenzioso di allarme che proviene dal popolo nei confronti del ceto dirigente. Non solo, ma la questione della qualità etica della pubblica amministrazione, oltre che della politica, è la condizione del funzionamento delle istituzioni e della bontà e concretezza di qualunque riforma istituzionale. In questi giorni siamo "allagati", negli elzeviri e nelle cronache politiche, dal dibattito sulle riforme costituzionali e istituzionali, starei per dire stucchevolmente: potrei forse sintetizzare questo balletto con «io do un'ammuina di premierato a te, tu dai una riformella elettorale a me, noi diamo un senatuccio delle Regioni a loro». Non è questo che si aspetta l'opinione pubblica. Si fa spesso involontaria o volontaria confusione tra i costumi privati e l'etica pubblica, non c'è dubbio, e già questa confusione è un dato devastante nel rapporto con l'opinione pubblica; questo decantato e sottolineato crollo delle ideologie, che è una verità, lascia capire che a questo crollo si sostituisce spesso il rischio del dominio dei poteri forti, l'istinto degli egoismi e anche una sorta di perversa religione del pragmatismo e dell'avventurismo furbastri. Meno Stato? Può darsi; io mi permetto di dire: più senso dello Stato.

ma per chi sente un po' di *pathos*, in particolare su questi argomenti, dovrebbero rappresentare degli impegni forti che reciprocamente ci indirizziamo, e li indirizziamo all'Esecutivo. Ebbene, nel documento, modestissimo, che a nome del Gruppo ho cercato di articolare, in effetti i punti sono di per sé concreti: stimolare ogni azione volta a prevenire, reprimere, sanzionare, accertare, confrontandosi con il comportamento medio - starei per dire - del cittadino onesto, perché è questo il parametro che noi dobbiamo adottare. Certo, nella nostra mozione non si manca di sottolineare gli importanti risultati ottenuti e anche l'impegno programmatico che il nostro Gruppo come programma elettorale ha declinato agli elettori. Io l'ho inteso così, e non da oggi: starei per dire, dal 1994; e e se non c'è questo spirito di porre l'etica pubblica al centro, viene meno la premessa di tutto il resto. Si sottolineano in questo documento i costi della corruttela e del malcostume, che alla fine vengono pagati dai cittadini; non si ignora il fenomeno di una corruttela diffusa, fenomeno che ho visto rispecchiato anche in altre mozioni di altri Gruppi. In sostanza, è giusto fustigare se stessi e i gangli della pubblica amministrazione, ma non ignorare quella corruttela o quella acquiescenza alla corruttela che in molte pieghe e in molti ambienti della società rischia di diffondersi. Si esprime un sostegno a quelle parti più attive e concludenti delle magistrature e delle forze dell'ordine che stanno pur collezionando importanti risultati su questo fronte. non riguarda solo il ceto politico, ma anche quello dei cosiddetti manager, di coloro che amministrano potentati, risorse e ricchezze ben superiori a quelle che il ceto politico si trovi ad amministrare. Si sottolinea - questo forse a differenza di altri documenti - la necessità del rispetto dell'equilibrio tra i diritti soggettivi della persona, che debbono essere tutelati e garantiti in un moderno e libero Stato di diritto, e la lotta agli abusi. Si richiama la doverosa attuazione delle convenzioni internazionali che la nostra Nazione ha sottoscritto e alla quale dunque è tenuta a dare concreta attuazione e rispetto alla quale, ormai da da molti anni - non riguarda solo questa breve parte di legislatura - siamo molte volte poco adempienti. Ancora un richiamo forte e articolato - al quale rimando per brevità - all'annunciato Piano nazionale anticorruzione, che va dai monitoraggi, dai controlli incrociati, dalla circuitazione dei dati, dal controllo di ogni singolo cittadino anche giovandosi della moderna informatica su ogni gara, appalto o realizzazione di opera pubblica. È molto importante che si dia seguito a questi impegni e a questi punti che sono declinati nel Piano nazionale anticorruzione, sul quale vigileremo anche come maggioranza rispetto alla forza, alla capacità e alla coerenza di attuazione. ricordo la inibizione alle candidature, alle cariche, agli incarichi di tutti coloro che siano condannati per reati contro la pubblica amministrazione; il richiamo alla semplificazione legislativa, perché non possiamo ignorare realisticamente che che molte volte anche la corruttela o la non schiettezza dei comportamenti è originata - non voglio dire costretta - anche da un intreccio di normative e percorsi che rendono la vita difficile a chi voglia onestamente operare; la necessità di una forte campagna nazionale di informazione e di sensibilizzazione al Paese intero, all'opinione pubblica, alle nuove e alle meno nuove generazioni.

Dobbiamo dimostrare con comportamenti ed esempi concreti, esigendo risarcimenti da chi fa danni, la realtà delle sanzioni, la premialità per chi denuncia e chi aiuta a scoprire le corruttele. Dovremmo segnalare all'opinione pubblica che è pagante questo piacere dell'onestà. Onorevole Presidente e onorevoli senatori, le norme sono importanti, certamente indispensabili e doverose, ma più delle norme vale restaurare un clima di rigore nell'etica pubblica, che deve essere pervasivo di tutti i livelli, sia decisionali che esecutivi.

Noi dobbiamo passare dal rispetto, quando c'è - e non sempre c'è - delle forme, al rispetto della sostanza, di quello che ho chiamato il clima dell'integrità e dell'etica pubblica, che rischiarano, motivano e rendono efficace ogni norma. Questo è lo spirito, al di là dei singoli commi e dei singoli passaggi, della nostra mozione e su questo terreno siamo pronti, perché è un dovere farlo,

Dall'analisi dell'area politica di appartenenza risulta emergere come la corruzione sia una realtà riconosciuta in maniera trasversale, da destra a sinistra, in tutto l'arco costituzionale.

di quegli amministratori che approfittano del loro ruolo di pubblico amministratore e approfittano del potere conferitogli dai cittadini, abusando chiaramente dei cittadini stessi che quel potere gli hanno In questi ultimi anni la domanda di comportamenti eticamente corretti e irreprensibili da parte degli amministratori pubblici costituisce un motivo lieto del dibattito politico del nostro Paese che, in coincidenza con l'emergere della tanto questione morale, ha avviato un processo di profonda trasformazione dell'assetto istituzionale. I casi di mala amministrazione, caratterizzati da vari tipi di accuse che vanno dall'abuso di ufficio, alla corruzione, alla concussione a carico di amministratori e politici

I numeri sono rilevanti: il Ministero della funzione pubblica ha presentato la relazione al Parlamento a novembre dello scorso anno (quindi è un fatto molto recente) e dai dati della cosiddetta mappatura sulla corruzione si evince come la mala amministrazione provochi tra corruzione, tangenti, frodi comunitarie e altre tipologie di reati danni per oltre due miliardi di euro; dati che non sono sicuramente frutto di fantasia, ma dati accertati dalla Guardia di finanza. Questo fenomeno porta sicuramente a una disaffezione del cittadino nei confronti della politica e prende piede e diventa non non solo prassi ma consuetudine l'equazione secondo la quale il politico è sostanzialmente una persona corrotta. I cittadini sono stanchi, stufi, fortemente amareggiati di vedere che i propri amministratori si comportano spesso in maniera scorretta. E questo possiamo tranquillamente affermarlo noi della Lega Nord, pur coscienti del fatto che è difficile trovare una composizione politica che possa tranquillamente scagliare la famosa prima pietra. Almeno fino ad Almeno fino ad oggi il nostro movimento può ritenersi abbastanza immune da questo fenomeno. Il tema è sicuramente molto complesso ed articolato - di questo siamo coscienti - e affrontarlo è sicuramente ma dobbiamo farlo con un atteggiamento positivo e propositivo, evitando il ricorso a demagogie o a soluzioni semplicistiche, che spesso rischiano di rimuovere i sintomi senza curare alla radice il problema. Anche Anche l'Unione europea ha evidenziato la natura spesso emotiva della legislazione anticorruzione, sottolineando come negli Stati membri dell'Unione tali interventi si siano sviluppati principalmente come reazione a casi specifici di corruzione o di comportamento spesso non etico; qualcosa di importante su questo argomento il Governo sicuramente lo ha fatto e lo sta facendo. Il 10 marzo del corrente anno il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", le cui proposte riguardano, in particolare, l'adozione di un Piano nazionale anticorruzione e la creazione di un osservatorio sulla corruzione, l'istituzione di una banca dati dei lavori pubblici e la promozione della trasparenza, con l'utilizzo spinto delle nuove tecnologie. Obiettivo centrale del provvedimento è rendere virtuoso il comportamento della pubblica amministrazione e sanzionare chi vìola la legge. Particolarmente significativo appare l'approccio al tema della corruzione, come informa il disegno di legge governativo, che non si limita a focalizzare l'attenzione sull'aspetto sanzionatorio e repressivo, ma punta sulla promozione dell'efficienza della pubblica amministrazione (cosa sicuramente apprezzata dai cittadini) quale primo strumento di prevenzione dei fenomeni di corruzione. evidente quindi che è necessario proseguire sul cammino di semplificazione dell'assetto amministrativo, già efficacemente avviato da questa maggioranza e attuato dal nostro ministro Calderoli, incentrando tale processo di riforma sul principio di sussidiarietà, che porta le decisioni più vicine al cittadino, consentendo a quest'ultimo più stringenti poteri di controllo nei confronti di noi politici. Sul piano politico il contrasto alla corruzione non può essere visto al di fuori del processo di attuazione del federalismo fiscale avviato dalla legge medesima. I fenomeni di corruzione della pubblica amministrazione si traducono infatti di regola (in maniera ora più indiretta ora più mediata, a seconda dei casi) in una lesione dell'efficienza della macchina amministrativa e, quindi, in un danno patrimoniale a carico della collettività. La corruzione, sia dei rappresentanti politici che dei burocrati, produce un cattivo funzionamento della pubblica amministrazione, sottraendo risorse ai cittadini stessi, ma soprattutto produce inefficienza dovuta all'incremento del costo dei servizi. Chiaramente, un servizio potrebbe costare di meno se non fosse gravato dai costi della corruzione. Se fino ad oggi si sono potute perpetrare pratiche contrarie al principio della buona amministrazione, tale situazione appare in larga misura imputabile alla mancanza di criteri e di procedure di valutazione delle politiche politiche pubbliche, in grado di misurare l'efficienza dell'operato degli amministratori, evidenziando scostamenti rispetto alla gestione standard. L'attuazione della legge sul federalismo fiscale, con il superamento del tradizionale, ma devastante, criterio della spesa storica e l'introduzione di percorsi obbligati che reimpostano la spesa pubblica sulla base di criteri standard, sembra destinata a offrire un contributo sicuramente determinante nella prevenzione dei fenomeni di corruzione. Con questa mozione, il nostro movimento chiede quindi al Governo di considerare come punto di partenza per un discorso mirato al tema della corruzione nella pubblica amministrazione il disegno di legge approvato il 10 marzo di quest'anno dal Consiglio dei ministri, di proseguire nel cammino di semplificazione della pubblica amministrazione avviato dall' inizio della legislatura ad oggi, con l'intento di ridurre quelle duplicazioni di funzioni e quelle sovrapposizioni di competenze che ostacolano una chiara identificazione delle responsabilità gestionali, introducendo il semplice ma efficace criterio di chi fa cosa, rendendo maggiormente lineari i processi decisionali, nell'ottica della trasparenza amministrativa verso i cittadini. Chiediamo inoltre di considerare prioritaria, anche ai fini del contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione, l'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, identificando nella definizione dei costi standard un efficace ma basilare strumento di misurazione dell'efficienza delle amministrazioni delle amministrazioni pubbliche e quindi dei politici stessi. Chiediamo infine di applicare, nel periodo della transizione dal criterio della spesa storica a quello dei costi standard, dei criteri premiali destinati ad incentivare quelle amministrazioni che, attraverso comportamenti virtuosi e l'attivazione di controlli interni, sappiano adottare efficaci politiche di prevenzione e contrasto della corruzione dei propri dipendenti.

mi limito soltanto ad illustrare la mozione a prima firma del senatore Rutelli per parole chiave. Mi domando in primo luogo se si possa riflettere sul significato primo della parola corruzione.

perché è qualcosa di più della mancanza di tornaconto per la pubblica amministrazione, è qualcosa di più del fatto che si rende inefficace la pubblica amministrazione: è il disfacimento dell'appartenenza, il disfacimento della comunità. Non è un caso che luoghi in cui la corruzione è perpetrata in maniera sistematica sono poi quelli in cui certamente la civiltà ha anche subito un brutto colpo.

il costume del Paese dei navigatori, degli inventori e dei santi sembra diventato il costume dei furbi e la furbizia e l'illegalità, quella microillegalità diffusa, sono le ancelle della corruzione, fanno strada. Questo è un costume che credo abbia qualche radice lontana e che non si debba guardare soltanto a logiche e comportamenti profondamente sbagliati di chi magari ha la responsabilità di dare di dare degli esempi, tenuto conto che c'è stato un tempo, non troppo buono per il Paese, in cui non si poteva neppure parlare di Patria, non si poteva parlare di merito, e dentro una scuola che non produce merito e dentro un'appartenenza che si vergogna di sé è difficile poi trovare il clima positivo e il senso profondo dell'appartenenza. Questa è la presa d'atto, e poi qualche considerazione. Ci sono così tanti cittadini con sentimenti forti di lealtà verso l'interesse generale, e talvolta sono frustrati nel valutare come il quadro normativo, che sembra sempre così ricco, alla fine diventa inefficace perché gli episodi di corruzione sono sempre snocciolati e sembrano non tramontare mai. La rassegnazione è un brutto segnale per una civiltà. Qualche parola chiave anche nell'impegno che si chiede al Governo. Anch'io personalmente sono convinto che le norme non possono essere tutto: non esiste norma alcuna che possa dare la cifra morale di una persona

allora che chiedere con insistenza al Governo l'attuazione piena ed integrale della Convenzione dell'ONU, per essere virtuosi dentro un sistema virtuoso più grande di noi, per non essere mai soli, la necessità che il vincolo virtuoso faccia sentire l'appartenenza ad una comunità più grande, è già a mio avviso un aiuto.

e credo che vada preso in considerazione anche l'annullamento di alcuni benefìci di legge quando intervengono reati di carattere economico nei confronti di una pubblica amministrazione. un reato contro la pubblica amministrazione è contro la comunità e l'appartenenza; è come rubare in chiesa. motivo, bisognerebbe stare significativamente attenti agli atti di furbizia che educano al contrario. Forse occorrerebbe rendere più efficiente l'azione della Corte dei conti

Io sono stato eletto all'opposizione, ma sono tra chi spera che il Governo del proprio Paese faccia bene; poi, magari potrò pensare dall'opposizione che noi potremmo fare meglio. Spero, comunque, che il Governo faccia bene; io tifo perché faccia bene! Su questo tema la speranza dei leali non può essere frustrata perché deludere una speranza è crudele ed illuderla è malvagio. Ritengo, pertanto, che il Governo al quale consegniamo questi suggerimenti potrebbe trovare utile - proprio perché è utile per il Paese che l'Esecutivo governi bene

per quasi tutti gli argomenti quando si tratta di illustrare e di discutere, per poi diventare piena soltanto al momento del voto,

bisogna dare atto ai colleghi di Italia dei Valori di avere assunto questa iniziativa per stimolare almeno in Parlamento un dibattito sul tema della corruzione, che sembrava agitare la politica italiana fino a qualche giorno prima delle elezioni regionali, in occasione di particolari circostanze e di iniziative giudiziarie, tanto da indurre il Governo, il 1° marzo scorso, ad annunciare l'adozione di un testo contro questo fenomeno criminale, che forse è tra quelli più gravi che possono colpire la vita delle istituzioni democratiche. Poi, come d'incanto, all'esito delle elezioni regionali, tale tema è scomparso dal dibattito politico e dal confronto,

che circoscriverebbe le politiche governative sulla materia alla fase dell'anticipazione di alcune norme sui controlli degli enti locali. Ora, io credo che questa iniziativa dell'Italia dei Valori e degli altri Gruppi dell'opposizione abbia un significato, perché cerca di indicare un preciso punto di chiarezza in Parlamento rispetto alle opinioni e rispetto ai fatti e agli atti che ciascuno di noi intende proporre sul tema. Non voglio dilungarmi su ciò che è stato già detto da altri colleghi e sui motivi di allarme che sono stati segnalati, così come non intendo soffermarmi neanche sull'analisi, diciamo così, sociologica del fenomeno, che potrebbe portarci fuori

parlamentare. Credo che per riuscire a fare una riflessione serena sulla questione dovremmo cercare di contenere al massimo la polemica e tentare in qualche modo di sviluppare un ragionamento che ci porti a produrre qualche risultato concreto, risultato che fino ad oggi non abbiamo avuto, e ad interrogarci sulla circostanza che forse questo sistema istituzionale, che ha diversi livelli territoriali di governo, ciascuno dei quali fuori controllo,

riflettere attentamente per comprendere che, al di là dell'esigenza di introdurre alcune disposizioni che adeguino il sistema e l'ordinamento

Oggi, nella cosiddetta democrazia bipolare dell'alternanza, in cui vi è un più veloce ricambio della classe dirigente e dei governi nazionali e locali

e nessuna può ritenersi o dichiararsi preventivamente immune dalla contaminazione di questo fenomeno. A qualsiasi livello territoriale di governo, e ancora di più a quei livelli che costituzionalmente hanno un maggior peso e un maggior potere,

come una società privata. In realtà, la privatizzazione dei servizi o di alcuni settori della pubblica amministrazione statale, regionale e locale, di fatto, ha prodotto la depenalizzazione di alcune condotte che erano considerate illecite. Oggi il concorso pubblico non è la regola ma l'eccezione, le assunzioni non le fa più la pubblica amministrazione ma le società miste, con regole che sono proprie del diritto privato ma non sono informate ad alcun criterio di trasparenza e ad alcun principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione; la selezione e la scelta del contraente, dei fornitori, degli appaltatori e quant'altro avviene secondo regole che sono quelle del diritto ma che non attengono ai principi costituzionali che regolano l'attività della pubblica amministrazione. Rispetto a tutto questo, che cosa è cambiato? È cambiato il titolo giuridico, ma la condotta che era illecita, tale era e tale resta sotto il profilo del suo disvalore morale, perché non vi perché non vi è alcuna distinzione tra il fatto che un soggetto venga assunto da una società per azioni privata interamente partecipata dal pubblico o da una pubblica amministrazione con criteri che non sono di imparzialità. Il problema è che un tempo quelle condotte potevano essere perseguite mentre oggi non sono più perseguibili. Dunque, c'è l'esigenza di adeguare l'ordinamento e di comprendere che non basta cancellare alcuni settori dell'amministrazione dello Stato o degli altri enti dal novero delle amministrazioni pubbliche per rimuovere o risolvere d'incanto il problema dell'utilizzo improprio delle risorse dei contribuenti italiani - di questo, infatti, si tratta - poiché questo è un fenomeno che nell'era dello pseudofederalismo trova una sua moltiplicazione, perché si sono moltiplicati anche i centri di spesa. È chiaro che tutta questa realtà ha bisogno di un adeguamento dal punto di vista ordinamentale, che deve essere introdotto e che noi - anche noi, ma non solo - con la nostra mozione tendiamo ad introdurre. Non parlo ovviamente delle delle altre ipotesi contenute nelle mozioni, perché non mi voglio dilungare su questi aspetti visto che, come diceva prima il collega senatore Gustavino, su tanti aspetti ci sono convergenze tra le varie mozioni, e dunque è inutile appesantire il dibattito da questo punto di vista. È chiaro che non basta solo questo: nella nostra mozione segnaliamo ad esempio la necessità che si costruisca un sistema di regole che prevenga i fenomeni di degenerazione. Tale sistema di regole deve certamente essere informato anche alla trasparenza dell'attività di ciascuno di noi.

che percepiscono ingenti retribuzioni per l'alto livello di professionalità che possiedono: il sistema di regole che riguarda la pubblicità e la trasparenza della consistenza patrimoniale e reddituale di questi soggetti è datato ed inadeguato, come dimostrano i fatti. fatti. Come parlamentare, ad esempio, ho l'obbligo di depositare la mia dichiarazione patrimoniale e la mia dichiarazione dei redditi e le eventuali

immunità parlamentari del Senato ha fatto un lavoro assolutamente pregevole da questo punto di vista, segnalando tutte quelle

perché è l'unico modo con cui possono scoprire la corruzione. A questo punto, debbo dire che quando ho sentito che che si riuniva il Consiglio dei ministri di questo Governo per iniziare una lotta seria alla corruzione sono rimasto stupito e ho ritenuto che finalmente si invertisse una tendenza. Non mi sono fatto le illusioni del collega Gustavino che ha sperato che questo Governo effettivamente mettesse in atto delle misure idonee a combattere la corruzione,

questo Senato. Ed è purtroppo la verità. Abbiamo detto che è un reato difficile, quasi impossibile, da scoprire. Che cosa stavamo discutendo stamattina in Commissione giustizia?

un'intercettazione di comunicazioni telefoniche occorrono evidenti indizi di colpevolezza per la corruzione - che deve essere anche indispensabile - si dice una cosa in contrasto

ma anche nel passato abbiamo fatto la stessa cosa. Cos'è che consente la corruzione? Ha ragione il quando dice che bisogna punire anche la corruzione privata, perché è diffusa; chiunque maneggia denaro pubblico, infatti, è suscettibile di essere corrotto,

finalizzata al finanziamento dei partiti politici, aveva come necessità fondamentale che ad essa partecipasse anche la burocrazia, era attraverso la burocrazia che si facevano i contratti di appalto, ed era attraverso la burocrazia che si riusciva a far assegnare gli che aveva finanziato i partiti e che aveva dato larghe adesioni (ed anche loro facevano la propria parte). Questa burocrazia, in gran parte, è lì, nei Comuni, nelle Province, negli enti pubblici, nelle società private, perché molte aziende di Stato e comunali sono state ridotte a società per azioni.

Come? Punendo severamente il falso in bilancio. Lo abbiamo fatto, lo ha detto prima il collega Li Gotti, per le società quotate in Borsa, addirittura

Per le altre società, quelle non quotate in Borsa, addirittura si è ridotto il reato: perseguibile a querela. Ma a querela di chi?

Mi volete dire, visto che di recente è venuto fuori in maniera evidente, come si possono fare quantità immense di soldi ai danni dello Stato e dei cittadini attraverso le cartiere, le cosiddette fatture false, se avete intenzione di fare qualcosa per rendere punibile immediatamente l'uso di fatture false senza aspettare che vengano impiegate poi nei bilanci? Io di tutto ciò non ho sentito parlare neanche nella vostra mozione: mozione: questo aspetto è saltato fuori nella riunione del 10 marzo del Consiglio dei ministri, di cui non si è saputo niente attraverso i giornali ma solo quello che ci avete detto oggi. Non c'è la lotta ai fondi neri; non c'è la lotta all'evasione fiscale, attraverso la quale si creano i fondi neri, né c'è la lotta alle cartiere,

È questo che dobbiamo tenere in grande conto. La Lega Nord ha parlato di lotta alla corruzione che il federalismo fiscale Ma perché, adesso che non c'è il federalismo fiscale in sede nazionale, in Parlamento, forse condanniamo e mettiamo all'indice chi ruba il denaro pubblico?

il principio fondamentale enunciato dalla nostra Costituzione sulla presunzione di non colpevolezza fino al passaggio in giudicato

questo accade - lo abbiamo visto anche di recente - nell'immediato non si parla di assoluzione per corruzione e di una sconfitta della giustizia nella lotta alla corruzione, ma si dice che l'imputato è stato perseguito ingiustamente dalla magistratura ed è stato assolto.

Senatore D'Ambrosio, la corruzione si combatte facendo il proprio dovere: lei fa il suo, io devo fare il mio. D'AMBROSIO *(PD)*. Si fa anche condannandola moralmente.

morale. Presidente, sono stupita del fatto che questa sera siamo riuniti in 20 persone. Stiamo toccando uno dei problemi più seri che abbiamo in questo momento nella società italiana, il problema della corruzione,

nel momento in cui si parla di questioni gravissime per il Paese, per l'economia, per l'occupazione, per i giovani e di problemi ordinari della giustizia siamo riuniti in pochissime persone. Questo non è uno spettacolo bello da dare a una scolaresca che è presente, perciò sono contenta che abbia assistito alla lezione del senatore D'Ambrosio. non posso che riportarmi a quanto il senatore D'Ambrosio ha già detto. Effettivamente non possiamo fare a meno di valutare ciò che è accaduto dopo che

la politica non ha approfittato di questa occasione, lasciando ancora una volta nelle mani del giudiziario la lotta contro la corruzione. Tutto questo è stato accompagnato da strumenti che contrastano un'effettiva volontà di combattere la corruzione. Mi riferisco innanzitutto al regime della prescrizione: cosiddetta legge *ex* Cirielli del 2005 interviene riducendo i tempi di prescrizione, facendo aumentare il numero di reati da dichiarare estinti e, quindi, i processi da vanificare, facendo inoltre decorrere il tempo della prescrizione separatamente per ciascuna delle prestazioni di denaro illecitamente percepite, con ricadute in termini di effettiva perseguibilità dell'intero illecito commesso in ambito corruttivo. che si comincia a far decorrere il tempo dall'ultima tangente. Si è abolita anche la figura del reato continuato. Quanto al falso in bilancio, credo sia dimostrato da tutti coloro che di questa materia si sono occupati (anche io, e non lo rinnego, me ne sono occupata nella mia precedente attività di magistrato)

recuperano attraverso il trucco dei bilanci e comunque la creazione di disponibilità extracontabili. Purtroppo - come dicevano anche coloro che mi hanno preceduto - dal 16 aprile 2002 è operativa la riforma degli illeciti penali amministrativi delle società commerciali, commerciali (decreto legislativo n. 61 del 2002), in conseguenza delle quali sono state ridotte le pene per il falso in bilancio e dunque aumentata la possibilità di estinzione del reato per prescrizione, con lo stesso decreto legislativo, inoltre, sono state introdotte soglie di non punibilità altissime, dando luogo ad una sorta di impunità che si potrebbe definire per modica quantità di fondi neri. Soprattutto per le società non quotate, il reato è stato reso perseguibile a querela delle parti offese quindi dovrebbero essere creditori o azionisti a querela da presentare contro gli amministratori. Naturalmente la perseguibilità del reato - lo voglio dire fino in fondo - è resa assolutamente improbabile in quanto non si è mai visto che un processo per falso in bilancio sia scaturito dalla denunzia del socio di maggioranza, che di solito è il mandante oppure il beneficiario del reato; perché è prevedibile che un socio di minoranza venga risarcito subito dopo aver subito il danno in modo che non presenti querela oppure che la ritiri, ed essendo facilmente ipotizzabile che il creditore, che è l'unico che potrebbe avere un effettivo interesse a querelare e far proseguire un processo, non sia a conoscenza della falsità dei bilanci. Devo rilevare che anche la riforma dei reati fiscali del 2000 ha prodotto un ulteriore danno poiché viene punito l'uso di fatture per operazioni inesistenti solo se superano una determinata soglia o se si riverberano sulla dichiarazione dei redditi. Questo Questo comporta che possono essere portate spese gonfiate o inventate tra i costi non deducibili e non tra quelli detraibili, in maniera da ottenere risorse fuori bilancio che servono per pagare tangenti, senza più commettere reato. Infine, il riciclaggio e l'autoriciclaggio costituiscono i principali canali di impiego dei proventi delittuosi, in particolare del crimine organizzato e dei reati contro la pubblica amministrazione, ma malgrado questo l'autoriciclaggio attualmente non assurge ad illecito penale e il Parlamento non ha ancora approvato i disegni di legge che sono stati proposti in materia dal Partito Democratico, come dalle altre opposizioni, procedendo ad una necessaria integrazione della normativa italiana in maniera da mettersi in linea con le legislazioni di altri Paesi e le direttive europee ed in maniera da consentire una collaborazione seria nella fase dei rapporti internazionali quando le autorità giudiziarie ricercano i fondi e li vogliono effettivamente sequestrare. sequestrare. In questo senso è anche assolutamente indispensabile che nel Paese sia rafforzata l'azione della magistratura contabile, rispetto alla quale va garantita l'assoluta ed effettiva indipendenza da altri poteri dello Stato. Invece questa indipendenza e questa azione efficace della magistratura contabile sono state gravemente pregiudicate dalle recenti riforme legislative, tra cui quelle che fanno capo ai decreti-legge 1° luglio 2009, n. 78, e 3 agosto 2009, che all'articolo 11, oltre ad indebolire sensibilmente le prerogative e i poteri della Corte dei conti, ne pregiudica in maniera rilevante l'indipendenza. Tutti ricorderanno il dibattito che abbiamo fatto sul cosiddetto processo breve. hanno avuto modo di inserire altre norme che indeboliscono l'azione della magistratura contabile e quindi la possibilità di ottenere risarcimenti di danni per la parte offesa, che è lo Stato; addirittura a carattere retroattivo. Signor Presidente, so che sto abusando del tempo a disposizione, ma penso che se vogliamo fare seriamente qualcosa di costruttivo dobbiamo avere il coraggio di analizzare quali sono stati gli interventi

la possibilità di combattere questo illecito così grave nelle sedi giudiziarie, addirittura indebolendo lo strumento delle intercettazioni o affievolendo altri strumenti che sono a disposizione, credo che difficilmente potremo fare un'opera seria per il Paese. È l'opera che noi legislatori siamo obbligati a fare, perché paradossalmente non solo non stiamo andando avanti, ma possibilmente stiamo andando indietro e questo è assolutamente inaccettabile. Per cui, al di là di tutte le buone intenzioni che si possono recepire nelle varie dichiarazioni di intenti, nei disegni di legge annunziati e mai visti del Governo, vorremmo che in concreto invece si attuassero

ad esempio - dimenticare che, nel recepimento della convenzione ONU contro la corruzione, non abbiamo voluto riproporre una autorità che deve occuparsi effettivamente di monitorare e contrastare il fenomeno, mentre abbiamo una autorità che comunque è posta nell'ambito del Governo

sia per carenza di strumenti sia per la posizione subordinata in cui si viene a trovare, di dare un quadro reale rispetto al quale il Governo e il Parlamento dovrebbero poi intervenire. *(Applausi

Purtroppo i numeri e le cifre confermano quanto sia dilagante il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione e quanto essa continui a dilagare. È evidente che questa piaga sociale trova nuova linfa nella certezza dell'impunità e nella assenza di controlli. I reati di corruzione sono gravi intanto perché denotano disprezzo verso coloro che hanno dato fiducia per svolgere una funzione pubblica, ma soprattutto perché colpiscono l'intera comunità civile dello Stato. Troviamo la conferma nel fatto che l'Italia, nella classifica mondiale, si pone in una posizione molto arretrata e soprattutto lontana dai Paesi più industrializzati tra i quali ci vantiamo di essere. Il fenomeno della corruzione è allarmante e occorrono provvedimenti concreti ed efficaci per affrontare questa lotta che ‑ ripeto ‑ è di civiltà. Ad oggi, credo che il Governo sia fermo all'annuncio mediatico. É una lotta da affrontare con strumenti idonei ed adeguati, con la coerenza e la determinazione di chi è convinto di volerla affrontare e di credere in un risultato. Non devono essere presi assolutamente in considerazione provvedimenti che in qualsiasi modo possono danneggiare la perseguibilità di questi reati. Non possono essere affrontate questioni quali quelle proposte nei disegni di legge sul processo breve o addirittura sulla limitazione delle intercettazioni telefoniche, se non si ha poi la certezza che l'introduzione di nuove norme vada nel senso dell'eliminazione di questo preoccupante fenomeno. Non si tralasci comunque l'aspetto fiscale. Non è da sottovalutare che la lotta all'evasione fiscale porta a scoprire intricati e complessi sistemi di finanziamento del malaffare ed è in questo che certamente rientra la corruzione e, di conseguenza, i perversi legami tra malaffare e mala politica. e concussione sono aumentati notevolmente ed è triste dirlo, perché - per chi come me ha lavorato in sanità - questi sono i settori più interessati. È certamente l'enorme mole di finanziamenti che rende in qualche modo vulnerabile il settore della sanità. La Corte dei conti sostiene che la sanità è «terreno fertile per comportamenti truffaldini o comunque per forme di sperpero di pubbliche risorse». Sono molte le tipologie di illecito segnalate: dagli incarichi illegittimi (come sosteneva il senatore D'Alia) al personale estraneo alle aziende sanitarie, ai doppi compensi percepiti dai medici fino alle irregolarità sulla esenzione dai ticket, oppure alla doppia o fraudolenta fatturazione della spesa. Per non parlare, poi, del sistema di gestione di beni e servizi, ove ci troviamo al cospetto di interessi di *lobby*. È assurdo, tanto per fare un esempio, che uno strumento medicale venga a costare alla sanità pubblica molto di più di quanto costi È necessaria, quindi, una serie rete di controlli, ma anche più trasparenza, perché è anche impensabile che i costi per beni e servizi siano tanto differenziati tra Regione e Regione. Ma, prima dei controlli, deve esserci la prevenzione. Ed è la stessa Corte dei conti ad auspicare che da parte della pubblica amministrazione ci sia «un uso delle risorse pubbliche che sia non solo legittimo, ma anche pienamente rispondente ai criteri di sana amministrazione» ovvero che produca «il migliore risultato possibile in termini di economicità e di efficacia». Questo è il vero problema: occorre combattere la corruzione, ad ogni livello, sia tra gli amministratori pubblici, sia tra i soggetti titolari di cariche elettive e di Governo. Combattere la corruzione è un obbligo dello Stato e questo Paese deve recuperare l'immagine che ha perso. È una questione di etica, molto sentita dal cittadino e inoltre rimane un grave costo che pesa sicuramente su tutta la collettività.

è già stato dimostrato abbastanza da questo dibattito e dagli interventi svolti dai colleghi che mi hanno preceduto come la questione della corruzione sia arrivata ad una diffusione e a una penetrazione che ormai sono dimostrate oltre ogni ragionevole evidenza. La condizione italiana, sotto questo profilo, è molto diversa dallo standard normale degli altri Paesi civili più avanzati e anche di quelli meno avanzati. La posizione dell'Italia nelle classifiche economiche svetta all'interno dei primi dieci, con qualche incertezza a seconda dei settori di cui si ragioni. Ma se se si va a vedere la posizione dell'Italia nelle classifiche del giudizio sulla corruzione od anche sulla libertà di informazione, noi scendiamo a posizioni lontanissime dal consesso dei Paesi civili. C'è qualche cosa che lede in modo intimo quell'immagine luminosa che l'Italia proietta di sé quando si ragiona in termini di cultura, di arte, di paesaggio, perfino di ricerca scientifica. Benché non vengano mai dati soldi alla ricerca scientifica, può capitare che l'Italia assuma delle posizioni pioneristiche, perlomeno su certi argomenti. Colpisce questo fatto. L'Italia di Abbado e di Pollini, per citare soltanto dei musicisti (perché non posso elencare troppi soggetti), è tradita

1.000 euro a testa, cifra che grava sulle spalle del cittadino italiano per un fenomeno che sembra invincibile, radicatissimo, ramificatissimo.

la competizione del merito, la competizione alla pari, la concorrenza. La corruzione svia le forze naturali dell'economia dal loro compito, le intercetta, le ferma e fa avanzare dei protagonisti opachi, di cui non si sa

Vorrei dire di più. In questa lesione della competizione alla pari, la corruzione è una sorta di azione determinata contro l'uguaglianza, proprio perché impedisce l'esercizio del confronto economico sulla base dell'eguaglianza. La corruzione appare come una sorta di tessuto invisibile che invalida e sostituisce la rete delle relazioni pubbliche che vengono condotte nella legalità. E' un altro mondo, un mondo parallelo, incisivo, che riesce a determinare anche la vita dell'economia legale. Non si sa più nemmeno quale sia il confine tra economia legale e economia

questo tipo di corruzione, che incide dentro e contro l'economia contro l'uguaglianza non è messa in atto da soggetti qualsiasi.

dell'amministrazione, del circuito degli affari, della stessa rappresentanza politica e che agiscono perlomeno in ogni caso all'interno della rete che è rappresentata dalla complessità delle relazioni di potere. Per dirla con una frase un po' sbrigativa, la corruzione è un'attività intima di una quota significativa, o in ogni caso non trascurabile, delle classi dirigenti. La corruzione non è

appaiono anche le figure devianti. I malavitosi appaiono dentro la prassi corruttiva, ma unicamente come strutture di servizio, come membri ausiliari e ancillari. Questo perché

in quanto tale dovrebbe essere affrontato. che anche le attività dell'attuale Presidente del Consiglio affondano in una realtà corruttiva purtroppo oramai chiaramente dimostrata, a onta del fatto che magari sotto il profilo giudiziario le cose siano state annebbiate. Ma voglio ricordare, ad esempio, il premio in miliardi che Craxi si è preso per la legge Mammì, che ha favorito, in maniera spudorata, un monopolio della comunicazione privata che in nessun altro Paese del mondo sarebbe stato tollerato. Anche nella vicenda Mondadori, nella vicenda Mondadori, c'è un sodale del Presidente del Consiglio che è stato condannato in via definitiva per aver corrotto un magistrato per far ottenere all'impresa del Presidente del Consiglio il possesso della più grande e, in un certo senso, classica

del Consiglio attuale sta anche la legislazione sul falso in bilancio. Il falso in bilancio, come è stato giustamente ricordato dei colleghi, ha una funzione specifica e produttiva dentro la costruzione corruttiva perché rappresenta il momento in cui si mettono da parte i fondi neri che devono essere utilizzati per corrompere. Ebbene, esso è stato reso un reato bagatellare e poco ci manca che costituisca oggi un titolo di premio. Siamo imbarazzati di fronte a questo, e in realtà dovremmo procedere in modo completamente opposto, ma in realtà non stiamo procedendo in modo completamente opposto perché, come è stato già ricordato, è stato soppresso soppresso l'Alto commissariato contro la corruzione e, soprattutto, le manovre in atto e, purtroppo, incombenti anche in questa Aula fanno pensare il peggio. Non sto a ripetere i concetti espressi, molto meglio di me, dai colleghi D'Ambrosio e Della Monica, ma la questione del processo breve è probante e, ancora di più, lo sono i passi minacciosi del provvedimento sulle intercettazioni. Se noi vogliamo affermare che lottiamo contro la corruzione non possiamo costruire un costruire un provvedimento legislativo che, in buona sostanza, tronca, in modo pressoché definitivo, la possibilità di indagare sui fatti corruttivi, in quanto priva i magistrati inquirenti di uno degli strumenti fondamentali.

quest'Aula si appresta a varare un provvedimento che, sostanzialmente, rappresenta il via libera per fare tutto ciò che è inconfessabile e non dicibile perché, ormai, tutto ciò che non è dicibile e non confessabile non verrà più conosciuto da nessuno. L'ignoranza calerà sull'opinione pubblica critica. La non conoscenza ci schiaccerà. Saremo costretti a parlare sotto voce di cose che sappiamo esistere ma di cui non possiamo più parlare perché ci sarà impedito di farlo. Noi siamo ad un passo gravissimo dell'evoluzione pseudodemocratica di questo Paese. Se poi si pensa che il soggetto che unisce questo passato di natura corruttiva alla prassi contro la corruzione di oggi si prospetta addirittura, in modo assolutamente sfacciato ed inaccettabile, come *dominus*

contro tale visione della riduzione della pluralità dei poteri ad un potere unico intestato ad una persona unica, noi ci batteremo fino all'ultimo. E ce la faremo, perché è un qualcosa di intollerabile per la democrazia italiana.

Signor Presidente, signori Sottosegretari, onorevoli senatori presenti, il fenomeno della corruzione, come già affermato da altri, non è solo questione di etica, seppur importante. È anche una questione economica, rilevante al punto tale che la pubblicistica parla di economia della corruzione o, meglio, di criminalità economica. L' economia della corruzione, difficile da accertare e misurare nella sua precisa entità, sembra che si attesti su valori molto alti. Il Servizio anticorruzione e trasparenza del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha stimato, solo per la pubblica amministrazione, un costo della corruzione pari a circa 60 miliardi di euro. Parliamo di una tassa occulta, pagata da ogni cittadino italiano nei diversi ambiti economici nei quali la corruzione genera effetti negativi. In particolare questa tassa occulta genera riduzione della crescita economica, deterioramento del meccanismo di funzionamento dei mercati e non attrazione degli investimenti esteri, inefficienza degli investimenti pubblici e inefficienza della distribuzione delle risorse. Proviamo a vedere questi aspetti con maggiore dettaglio. Per quanto riguarda la crescita economica, la Banca d'Italia ha mostrato che esiste un legame diretto tra questione morale e prosperità collettiva: dove maggiore è la corruzione, minore è il prodotto interno lordo *pro capite*. Viceversa, afferma sempre la Banca d'Italia, dove maggiori sono i comportamenti retti e virtuosi, maggiore è lo sviluppo della società: la probità, dunque, è una dote non solo per l'individuo ma per il Paese nel suo insieme. Anche la Corte dei conti ha affermato che «il fenomeno della corruzione è talmente rilevante e gravido di conseguenze da far più che temere che il suo impatto sociale possa incidere sullo sviluppo economico del Paese». Tirarsene fuori, quindi, è una necessità per la società nel suo complesso. Circa il deterioramento del funzionamento dei mercati, la corruzione agisce come un costo fisso che incide pesantemente nelle decisioni di investimento delle imprese aumentandone i prezzi. Essa produce, altresì, un fattore determinante per la non entrata e, spesso, per l'uscita dal mercato, soprattutto delle piccole e medie imprese che sono il nocciolo duro della nostra economia e che non hanno i mezzi strutturali e finanziari delle grandi imprese. Oltre a perdere competitività, i mercati corrotti non attraggono investimenti di capitale straniero e sono segnati da una bassa crescita (troppe barriere all'entrata, troppi rischi di investimento). Circa gli investimenti pubblici, in Italia è stata confermata una relazione positiva e significativa tra gli investimenti nel settore delle costruzioni e dei lavori pubblici, da un lato, e gli indici di corruzione e di criminalità organizzata, In questo contesto la corruzione ha l'effetto, sia di far lievitare la spesa per ogni opera finanziata, sia di distorcere l'allocazione delle risorse tra le opere da realizzare. La corruzione incide sull'offerta dei servizi pubblici imponendo un prezzo maggiore e una quantità inferiore di quanto si determinerebbe in assenza della stessa. Infine, per quanto riguarda la distribuzione delle risorse, la corruzione avvantaggia chi possiede i mezzi per ottenere benefici personali sopprimendo la meritocrazia e, per questa via, la gestione efficiente delle risorse. Combattere la corruzione è possibile ma servono azioni decisive. In particolare, occorre tutelare la competitività in tutti i settori, specialmente nel settore delle costruzioni e dei lavori pubblici. Occorre poi che la trasparenza sia associata ai meccanismi di competizione. È un bene da tutelare con cura se è vero, come ha affermato il presidente della Corte dei conti, che «laddove manca la trasparenza si genera il cono d'ombra entro il quale possono trovare spazio quei fatti di corruzione o concussione che rendono indispensabile l'intervento del giudice penale». Nel rapporto dei Paesi GRECO (Gruppo di Stati (Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa) si afferma che in Italia la corruzione ha assunto un carattere sistemico, in cui non vi è più la contrapposizione tra una società politica corrotta e una società civile sana ed onesta: al contrario, il sistema della corruzione si è radicato nella società, innervandosi in profondità nel mondo delle professioni, dell'imprenditoria e della finanza. I Paesi GRECO hanno inviato all'Italia 22 raccomandazioni riprese nella mozione del Gruppo del Partito Democratico. È necessario che esse, non più rinviabili, vengano accolte dal Governo nel nostro ordinamento. Ed è, altresì, necessario che il Governo investa nell'istruzione per costruire una società avversa alla corruzione. Esiste infatti una relazione negativa tra livello di istruzione e quello della corruzione: minore è l'istruzione, maggiore è la corruzione. Un alto livello di istruzione è associato ad una società più preparata e meno propensa a comportamenti corruttivi; cittadini più istruiti sono più consapevoli e informati e in grado di meglio scegliere una classe dirigente di livello morale elevato. L'aumento vertiginoso degli episodi di corruzione denunciati nell'arco di tempo che va dal 1992 al 1996 non deriva da un'impennata nella realizzazione di questo tipo di delittuosità, quanto invece dal fatto che la corruzione ad un certo punto è venuta alla luce, attraverso una brusca ed energica contrazione della cosiddetta cifra nera. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, la corruzione è presente nel nostro sistema economico da sempre; tuttavia, le vie per contrastarla efficacemente esistono e sono praticabili. Il miglior nemico della corruzione risiede, come dice il mio collega presidente Morando, in un costante ed efficace agire della politica che faccia della trasparenza il suo principale connotato. È dalla trasparenza dell'azione amministrativa che bisogna partire se si vuole combattere questo drammatico fenomeno con l'obiettivo di contrastarlo, prima, e sconfiggerlo, poi. Infine, signor Presidente, le affinità sul tema in discussione hanno portato i Gruppi del Partito Democratico e dell'UDC a convergere su un ordine del giorno comune, a firma dei senatori Finocchiaro, D'Alia, Zanda, Bianchi, Della Monica, Lusi e di altri senatori, che sostituisce le due mozioni presentate.

Leggo in alcune mozioni presentate che trasparenza nella pubblica amministrazione e lotta alla corruzione sono elementi che fanno parte dei programmi di governo di tutti gli

valori, perché si vanno a violare le sensibilità delle persone e delle coscienze; si producono - come abbiamo ascoltato - danni spesso irreparabili sul piano morale e materiale. Sicuramente sono più devastanti i primi dei secondi: il danno morale non investe solo chi si macchia di una colpa o - diciamolo francamente - di un reato, né coinvolge esclusivamente le categorie alle quali egli appartiene (il politico, l'amministratore, il *manager* infedele dell'azienda),

la tradizione di onestà, che non può che essere condivisa in una società. Per poche mele marce mettiamo a repentaglio queste sensibilità ed onestà condivise e diffuse. vi sono anche aspetti che si riferiscono al mandato politico, di cui noi siamo portatori. Si viene eletti da qualcuno e, quindi, chi corrompe o chi si lascia corrompere commette un autentico reato di tradimento (stavo per dire di alto tradimento, ma non vorrei esagerare): un tradimento nei confronti del mandato che ha ricevuto, della gente che gli ha dato la fiducia e della storia di tanti cittadini ai quali magari farebbe comodo rubare per aiutarsi a vivere meglio, ma non lo fanno perché non vogliono cadere in questo tipo di tradimento. Ecco perché oggi noi, qui, idealmente,

Allora noi abbiamo anche il dovere, in questo momento, visto che siamo portatori di un mandato parlamentare, di parlare a nome della gente, ma, almeno su questi temi, non con i toni e gli accenti paludati della politica, bensì con le parole forti,

il nostro rispetto). Qualcuno tra noi ha mantenuto quel salutare rapporto settimanale o quotidiano con la generalità dei cittadini, con i tesserati del proprio partito. Bene, quel tipo di esperienza aiuta perché ci consente di riscontrare ogni giorno i loro umori, di raccogliere i loro malumori come salutare lezione di vita prima ancora che come feroce e duro controllo democratico. La politica, quella con la «P» dei Palazzi, affronta questi temi con strumenti ispirati a prudenza che la gente non capisce, a tolleranze che la gente fa ancora più fatica non solo a capire ma ad accettare. La politica, quella della «P» dei Palazzi, lo fa con neologismi che si chiamano garantismo Io sono tormentatissimo di fronte a questi neologismi, princìpi condivisibili sul piano teorico e anche filosofico, se volete, ma ambigui e pericolosi per la loro indefinitezza,

perché è la gente che deve capire e non è solo nei tribunali che questi problemi vanno risolti. Ecco allora che io sarò grato a chiunque mi aiuti a capire che cosa significhi garantismo. garantismo. Sicuramente significa consentire a tutti coloro che sono accusati di qualcosa di avere la possibilità di difendersi e di dimostrare di essere estranei all'accusa, si chiede alla persona di farsi carico della responsabilità di dimostrarlo. Giustizialismo spesso suona come un'accusa nei confronti di chi chiede chiarezza e giustizia.

chi lo fa nell'esercizio di un mandato pubblico danneggia un intero sistema che non gli appartiene e del quale, in quel momento, egli si dimostra indegno. Condivido quindi, fra le conclusioni del collega Benedetti Valentini, ma non solo, ne ho sentite altre di colleghi di ogni schieramento, la proposta di escludere da qualsiasi tipo di candidatura o di mandato pubblico chi sia stato condannato per reati di corruzione o concussione.

e per qualsiasi incarico, senza eccezioni e non, per esempio, solo per cinque anni, come qualcuno aveva proposto, perché sarebbe un modo per prendere in giro la gente. Chi ha tradito lo Stato e i cittadini non può immaginare di tornare come nuovo dopo un certo periodo di tempo. di tempo. La favola di Biancaneve la racconto anch'io ai miei nipotini, ma non credo molto alla sua verginità, così come non credo alla verginità riconquistata di chi si è macchiato di questo genere di reati solo perché sono passati cinque anni. Infine, signor Presidente, mi chiedo se questo modo di ragionare sia giustizialista o garantista. Penso che sia le due cose insieme se noi spostiamo il significato di questi termini dal soggetto che tradisce a quello che viene tradito, cioè al cittadino, che merita di essere garantito nella sua integrità e merita di essere ascoltato quando chiede giustizia.

Grazie